della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Laura Bottici per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale

di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore, senatore Balboni, se intende intervenire.

ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti relativi a un procedimento penale per diffamazione col mezzo della stampa, originato da una querela sporta in data 21 gennaio 2019 dal signor Antonio Giudice nei confronti del senatore Stefano Candiani. Oggetto della querela è un comunicato stampa dell'allora Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Candiani, pubblicato il 15 gennaio 2019 sulla piattaforma Facebook, attraverso la pagina ufficiale «Lega Sicilia Salvini Premier», dal titolo: «Candiani risponde ai contestatori gelesi: "Felice di dare ai siciliani onesti la certezza di un partito fatto da persone leali e serie"». Tale comunicato, inoltrato agli organi di stampa e pubblicato anche da altri quotidiani *online*, conterrebbe, ad avviso del querelante, espressioni offensive e diffamanti nei suoi confronti. La Giunta ha ritenuto, come lei ricordava, che i contenuti dell'atto di sindacato ispettivo presentato in Senato dal Gruppo della Lega il 27 giugno 2019 siano idonei a far ritenere configurabile il nesso funzionale richiesto dalla Corte costituzionale per la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, essendoci una sostanziale corrispondenza contenutistica tra l'atto *intra moenia*, ossia la predetta interrogazione, e l'atto *extra moenia*, ossia la dichiarazione su Facebook. si fa anche presente che, in data 6 novembre 2020, il presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta copia degli atti di un procedimento civile nei confronti dello stesso senatore Candiani, trasmessi dal tribunale ordinario di Gela, vertente sui medesimi fatti oggetto del citato procedimento penale. Per una più analitica esposizione delle argomentazioni a base della deliberazione della Giunta, faccio comunque rinvio alla relazione scritta già depositata in Aula.

sulla quale tra l'altro ho votato a favore in Giunta, presentata dal relatore Paroli. Mi permetto soltanto di evidenziare all'Assemblea che, al di là delle considerazioni svolte dal senatore, qui siamo in presenza di una macroscopica insussistenza

Pertanto, a nostro modesto parere, il magistrato avrebbe dovuto archiviare questo procedimento e non trasmettere gli atti al Senato. Ragione per cui noi voteremo a favore della proposta del relatore Paroli.

illustrate dal relatore, senatore Paroli, ma anche l'intervento del senatore Balboni. Il caso del senatore Candiani merita particolare attenzione, perché forse è uno dei più emblematici, se non il

il numero delle procedure che andiamo oggi a verificare, soprattutto in tema di espressione di opinioni. Talvolta infatti, si formulano accuse nei confronti dei parlamentari senza

ripeto, è un caso emblematico che ci deve far riflettere e forse dovrebbe anche essere oggetto di una discussione, che peraltro in Giunta - lo voglio dire - abbiamo già affrontato. Annuncio pertanto il voto favorevole di Italia Viva alla proposta illustrata dal relatore, senatore Paroli.

Qualche riflessione mi viene suggerita dall'intervento del collega Balboni e ora dall'intervento del collega Cucca: in virtù delle pronunce ormai consolidate della Corte costituzionale, normalmente andiamo a verificare se nelle dichiarazioni rese *extra moenia* vi sia una corrispondenza di vario tipo con le dichiarazioni che vengono fatte in Aula. In questo caso, giustamente, siamo stati tutti, o quasi, d'accordo nel ritenere che non si può arrivare al punto di censurare una libera espressione non solo del diritto di critica, ma del ruolo stesso del parlamentare. Aggiungo che per esercitare per esercitare l'azione penale è evidente che non basta che ci sia qualcuno che si dica leso o offeso e questo ne è il classico caso. caso. Mi scuserà il collega Candiani se approfitto dell'argomento per dire che questo è proprio uno dei punti che noi proponiamo nella riforma del processo penale, nel senso che

deve essere ragionevolmente certa della possibilità che l'impianto accusatorio possa far giungere a una condanna. Ho approfittato di questo caso perché è uno tra i più sereni. mi perdonerà il collega, ma è esattamente uno di quei casi in cui pacificamente - e lo sarà ancora di più quando sarà approvata la riforma del processo penale - non verrà

Si tratta più che altro di opinioni espresse all'interno di una formazione politica, che nulla hanno a che vedere con il profilo della diffamazione, così come è stato già detto dal senatore Balboni e dal senatore Cucca. Quindi, dichiariamo

bisogna affermare che il reato ipotizzato dalla querela appare, nel caso di specie, manifestamente infondato. Anche restando nel solco delle attribuzioni costituzionali del Senato, il nesso funzionale tra l'atto *extra moenia* e l'atto *intra moenia* appare evidente e indubbio, con conseguente configurabilità della prerogativa. La dichiarazione oggetto della querela nel caso di specie si sostanzia in un comunicato stampa dell'allora sottosegretario di Stato al pubblicato nel gennaio 2019 sulla piattaforma Facebook, attraverso la pagina Lega Sicilia Salvini Premier, dal titolo «Il senatore Stefano Candiani risponde ai contestatori gelesi: "Felice di dare ai siciliani onesti la certezza di un partito fatto da persone leali e serie!"». Tali affermazioni rientrano nel naturale svolgimento del diritto di critica politica che costituisce il *proprium* della funzione parlamentare. Un parlamentare che non segnali situazioni di illegalità, che non denunci pubblicamente eventi illeciti verrebbe meno all'adempimento del proprio ruolo e delle proprie funzioni. Il diritto di critica politica è stato, nel caso di specie, esercitato anche attraverso un'interrogazione presentata dal Gruppo Lega nel giugno 2019, nella quale si denunciavano rilevanti situazioni di illegittimità nello svolgimento di attività politico-elettorali nei territori in questioni. La coincidenza contenutistica tra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia* nel caso di specie sussiste e anche il disallineamento temporale tra tali due atti non è idoneo a incidere in alcun modo sul nesso funzionale, quindi sulla prerogativa, la cui sussistenza è quindi palese. Preciso che la ragione del disallineamento temporale tra dichiarazione oggetto di querela (gennaio 2019) e atto di sindacato ispettivo (giugno 2019) è dovuto al fatto che in quel periodo il senatore Candiani era sottosegretario di Stato, e in quanto tale appariva del tutto inopportuno sotto il profilo della correttezza istituzionale che lo stesso presentasse atto di sindacato ispettivo in qualità di senatore. Sotto tale profilo appare evidente che la prerogativa della insindacabilità sussiste e che qualunque tesi contraria finirebbe per impattare sul ruolo politico e sulla funzione di denuncia pubblica intrinseca allo stesso, con uno svuotamento delle funzioni politiche e parlamentari pericoloso per la democrazia e anche per la legalità. I fenomeni di illegalità vanno denunciati pubblicamente e non nascosti, specie da chi abbia responsabilità politiche, e chi si sottrae a tale onere diventa in qualche modo complice dei fenomeni criminali che gli stessi determinano su vari piani, compreso quello dei brogli elettorali. La denuncia del senatore Candiani è coraggiosa, pienamente legittima e coperta dalla prerogativa della insindacabilità.

ha deliberato a maggioranza per l'insindacabilità, ma con il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. Sottolineo che da allora è trascorso

giacché, nel frattempo che qualsiasi decisione sarà presa qui oggi, il diritto alla giustizia è già stato compresso in attesa della nostra delibera. Quando sento dire in questa stessa Aula che è necessario abbreviare i tempi della giustizia, penso che in realtà non lo si voglia fare. Sono parole vuote, come quelle che ho finora parentesi - del mio Gruppo in Giunta, posso dire senza timore di smentita che il nostro obiettivo, tanto in Giunta quanto in Aula, è stato sempre studiare a fondo i casi, approfondire tutti gli aspetti, curando di assicurare le garanzie costituzionali in tutti quei casi in cui siano davvero in gioco i valori fondamentali della persona coinvolta, garantiti dal nostro quadro costituzionale e dalle carte internazionali. In proposito, apro un'altra parentesi. Voglio sottolineare

puntualmente e accuratamente evitato di nominare un membro del MoVimento 5 Stelle quale relatore di un qualsiasi caso.

Il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato della Repubblica deve dare una risposta. L'impegno c'è stato. In particolare, in materia di insindacabilità in Giunta l'attività del MoVimento 5 Stelle si è sempre basata su un'attenta disamina oggettiva, guardando alle situazioni specifiche, alle peculiarità, come - ad esempio - nel caso in esame. C'è una peculiarità - lo hanno detto in molti - e sembra che la querela derivi da una sorta di vendetta politica o da una ripicca per vicende politiche locali. Se c'è stata una vendetta politica - non lo metto in dubbio - ciò è ascrivibile ad altri argomenti e a disarmonie interne ai Gruppi politici, che appartengono a problematiche di tutt'altra natura natura da risolvere altrove tramite le normali tutele ordinamentali. Gli strumenti attualmente previsti per tutelare la libertà di espressione di ogni cittadino, che sia senatore o meno, esistono e sono e sono più che adeguate, tant'è che esprimere opinioni e critiche politiche oggi in Italia per fortuna non è assolutamente reato. Anche il relatore rileva l'insussistenza del reato, essendo evidente che il senatore Candiani in quell'occasione stava esercitando un semplice diritto di critica pienamente legittimo. allora, il senatore Candiani si è appellato all'insindacabilità e, soprattutto, perché noi dovremmo concederla? Vogliamo assecondare l'abitudine a un privilegio? Non sarebbe stato più opportuno

teniamo ben presente che, ogni qualvolta ci si appella all'insindacabilità prevista dalla Costituzione, si comprime il corrispondente diritto alla giustizia del cittadino e questo è grave. motivo per cui l'insindacabilità può valere solo quando si riscontra uno stretto nesso funzionale con l'attività parlamentare e non è allargabile a piacere per il solo fatto di essere parlamentari, con ciò facendola decadere decadere da tutela dell'indipendenza dei poteri dello Stato a odioso privilegio. Proprio per questo, il MoVimento 5 Stelle è l'unico a rinunciare sempre all'immunità.

sottolineare che ho analizzato i documenti e manca del tutto il requisito del legame temporale che avvalori il nesso funzionale con l'attività parlamentare. L'unica attività attinente riscontrata è un atto ispettivo depositato dalla Lega e solo annunciato dal senatore Candiani

e oggettivo sono completamente mancanti i requisiti necessari per concedere l'insindacabilità richiesta. Eppure, ci si benda gli occhi di fronte a tanta evidenza perché si vuole comunque sfruttare il privilegio di essere parlamentari e ciò è grave e sbagliato. Concludo ribadendo che uscire fuori dai limiti individuati dalla Corte costituzionale ha come unica conseguenza svilire le prerogative in questione, perché trasforma tutto in un privilegio personale e, quindi, in una sorta di impunità inaccettabile, mentre spetta alla magistratura ordinaria valutare la vicenda.

Prima di porre in votazione mi corre l'obbligo di ricordare che l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, non è

di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Candiani costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68,

Signor Presidente, la vicenda trae origine da alcune dichiarazioni rese dal senatore Giarrusso in una manifestazione pubblica tenutasi a Porto Empedocle il 31 marzo 2019. In quella occasione il senatore pronunciava alcune frasi ritenute diffamatorie dall'attore Filippo Caci, che lo ha citato in giudizio davanti al tribunale civile per chiedere il risarcimento del danno. Il senatore Giarrusso pronunciava la seguente frase: «Noi lo sappiamo chi ci sta dietro Caci e non lo sa soltanto Ida Carmina e i cittadini di Porto Empedocle. Lo sappiamo in Commissione antimafia, in Parlamento e al Governo». Come è noto, nel caso in cui una dichiarazione resa *extra moenia* possa integrare astrattamente l'ipotesi del reato di diffamazione, per giurisprudenza costante occorre, per invocare l'insindacabilità della stessa, una corrispondenza con attività parlamentare svolta *intra moenia*. Io richiamo integralmente la relazione, che è stata approvata a maggioranza dalla Giunta - come lei, Presidente, ha appena ricordato - per ricostruire l'attività parlamentare del senatore Giarrusso in materia di in materia di antimafia all'interno delle istituzioni del Senato e della Commissione antimafia; nonché per concludere che - ad avviso della Giunta e del sottoscritto relatore - esiste in questo caso un chiaro nesso funzionale che ci porta pertanto a proporre all'Assemblea l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giarrusso, nel caso che ci occupa,

non stiamo a fare la protezione di nessuno, ma ci dedichiamo ad applicare i precetti costituzionali, che sono in questo senso le prerogative dei parlamentari.

entrato in quest'Aula. Come bene ha esposto il senatore Balboni, ci troviamo in presenza di un caso abbastanza chiaro ed evidente.

possibilità mediatiche e dove le situazioni sono molto diverse da quelle che c'erano quando è stata scritta la Costituzione. Ci stiamo ponendo il tema di come possa essere tutelata in questa società molto mediatica e di grande sovraesposizione la presunzione di innocenza: ridiscutiamo giustamente che cosa è la cultura delle garanzie. esaminando è un caso che si colloca proprio su una linea di riflessione di confine perché certamente

politica che si può e si deve spingere anche alla denuncia politica. I Costituenti, che uscivano dal periodo del fascismo, hanno voluto tutelare questo: bene. Qui però,

Non si processano le persone a furor di popolo e non è che, siccome sei un parlamentare, tra l'altro componente della Commissione antimafia, puoi farlo o, meglio, se lo fai, te ne assumi le responsabilità e in un giudizio farai valere tutti quei criteri di critica, di opinione, di eccesso che la legge e la giurisprudenza consentono. Ciò che noi non possiamo consentire è dire che, siccome sei un parlamentare, puoi fare un processo in piazza,

Signor Presidente, la vicenda di cui stiamo trattando in questa sede nasce dal fatto che il querelante avrebbe ravvisato nelle parole pronunciate dal senatore Giarrusso la volontà di ingenerare nell'opinione pubblica l'idea distorta di uno svolgimento di attività politica, da parte del medesimo soggetto, in modo illegale, con presunte collusioni con la criminalità organizzata attraverso il riferimento, più o meno esplicito, con informazioni che il senatore deterrebbe in qualità di parlamentare e membro della Commissione antimafia. Il senatore Giarrusso, attraverso le memorie depositate, ha parlato di travisamento del discorso squisitamente politico in cui qualsiasi riferimento al querelante era puramente marginale rispetto al tema trattato, ossia dinamiche politiche afferenti al Comune di Porto Empedocle. Sul tema occorre rilevare come l'esercizio del diritto di critica politica deve essere oggetto di giudizio in ambito processuale, mentre alla Giunta spetta esclusivamente il compito di valutare la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità sulla base dei parametri e dei criteri enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ad avviso del mio Gruppo, mancano i predetti parametri, il nesso funzionale tra attività parlamentare e dichiarazioni *extra moenia* non sembra ravvisabile in una semplice promozione di una disposizione normativa alla legge di bilancio del 2019, che non si sostanzia né nella presentazione di un emendamento, né di un altro atto non avente natura legislativa precedente alle dichiarazioni rese. Inoltre, deve essere verificata l'effettiva mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal querelante e la tesi difensiva. Ciò può essere esclusivamente valutato in ambito processuale. Pertanto, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità e, quindi, esprimeremo un voto contrario alla relazione.

è stato sostanzialmente accusato dal senatore Giarrusso di svolgere la propria attività politica in modo illegale e con presunte collusioni con la criminalità organizzata. La frase che è stata pronunciata nel corso di una manifestazione di piazza a Porto Empedocle, il 31 marzo 2019, è molto indicativa,

di Porto Empedocle. In questo modo il senatore Giarrusso ha avallato il sospetto nell'opinione pubblica di possibili elementi investigativi dei quali il senatore sarebbe direttamente informato per il suo ruolo di parlamentare e membro della Commissione antimafia. Si è difeso dicendo che l'accenno a Caci è assolutamente marginale, mentre fa direttamente il nome di Caci - quindi non può essere marginale non risulta che in Commissione antimafia il signor Caci sia stato mai oggetto di attenzione. Pertanto non credo sussista la finalità divulgativa di attività parlamentare, proprio perché nell'attività parlamentare della Commissione antimafia il signor Caci non ha mai trovato alcuna collocazione, alcuna attenzione.

che sussista la insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giarrusso, coerentemente con quanto già votato in Giunta.

concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo

di deliberare che le dichiarazioni rese dalla senatrice Laura Bottici costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il fatto riguarda le opinioni espresse dalla senatrice Bottici nel corso di un'intervista rilasciata nel lontano settembre 2013 alle emittente locale TV News 24, in cui avrebbe offeso la reputazione degli amministratori e del sindaco di Carrara in merito ai loro rapporti con gli imprenditori del marmo e con riferimento alle indagini avviate dalla procura di Massa sulla cosiddetta evasione alle cave. La questione riguarda il contributo sull'estrazione dovuto al Comune di Carrara Grazie a un accordo firmato il 29 luglio 2009 dalle associazioni di categoria e dal Comune, tale valore venne fissato a una cifra inferiore all'effettivo valore di mercato producendo un vantaggio per gli imprenditori del marmo e un danno per le casse comunali. Nell'intervista oggetto di querela la senatrice Bottici ha pronunciato la seguente frase: «Nell'unico intervento che ho fatto in Senato su questo argomento ho dichiarato che spesso i rapporti tra l'amministrazione e gli imprenditori locali che si occupano di cave sono pseudo mafiosi - è questa la parola incriminata - questo vi dice come io posso pensarla sull'argomento». Dall'esame delle attività compiute dalla senatrice Bottici *intra moenia* è emersa non soltanto la sussistenza del nesso funzionale, perché di questi argomenti la senatrice Bottici si era già occupata nella sua attività istituzionale, ma addirittura la corrispondenza, quasi testuale,

la Giunta ha approvato, a maggioranza, di proporre all'Aula l'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Bottici ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Mi permetto di aggiungere, signor Presidente, che, da un attento esame della frase incriminata, ritengo che - anche in questo caso come nel caso del senatore Candiani - si sarebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere e la magistratura non avrebbe dovuto impegnare quest'Aula

Probabilmente la senatrice Bottici voleva dire para mafiosi, ma, in concreto, ha detto pseudo mafiosi. Manca, quindi, ogni offensività in tale affermazione. Ragion per cui vale la pena concludere per la insindacabilità. *(Applausi)*.

Viene il sospetto che voi abbiate voluto portare in Aula la questione sapendo che, comunque, ci sarebbero stati il centrodestra, il Partito

visto e considerato che, a differenza vostra, tra l'odio e il principio noi scegliamo il principio e scegliamo i valori. Questa è la nostra differenza!

Senatore Croatti, mi sembra che abbia espresso un'opinione.

Non si riesce a capire cosa dite e, quindi, è inutile che vi agitiate. Ognuno stia al proprio posto. Il Senatore Questore è intervenuto. Gli amici della Lega si accomodino. Ai senatori 5 Stelle dico che non è il loro turno di parlare. Ha parlato il senatore Romeo

prego, senatrice Ginetti. Signor Presidente, intanto vorrei dire che la Giunta, per ogni caso che è necessario istruire ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge un attento esame della documentazione, per analizzare i casi nel fatto e in diritto.

Spesso ci sono casi controversi, ma di certo altri sono anche più semplici, perché noi comunque dobbiamo seguire i principi della giurisprudenza che ci sono stati consegnati, in particolare dalla Corte costituzionale, con una serie di sentenze del 2014, del 2011 e anche del 2013, che ci indicano esattamente in che modo e quali principi dobbiamo andare a

abbassare il tono della voce per consentire alla senatrice Ginetti di essere ascoltata da chi lo desidera.

Rispetto al fatto che stiamo discutendo, ossia l'intervista rilasciata nel settembre 2013 all'emittente locale Ttnews 24 dalla senatrice Bottici, appare evidente l'esistenza di atti tipici interni della senatrice stessa, che ci permettono di verificare una corrispondenza sostanziale delle dichiarazioni rese e, quindi, di ritenere applicabile l'articolo 68, della Costituzione. Ricordiamo, anche in questo caso, che noi non stiamo analizzando un singolo caso per la tutela particolare e specifica della senatrice Bottici, ma ma stiamo compiendo un dovere costituzionale di tutela della democrazia, in riferimento all'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare; non solo di democrazia, ma soprattutto di autonomia nell'esercizio della funzione legislativa, politica, parlamentare, rispetto ad altri organi dello Stato. È una conquista che ci hanno consegnato i nostri Padri costituenti, i Padri fondatori della Repubblica democratica italiana, ai quali noi dobbiamo un tributo di ringraziamento. Per questo siamo chiamati ad analizzare ogni caso con molta attenzione,

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché credo che la collega Bottici rappresenti il vero spirito del MoVimento 5 Stelle. Tuttavia io non mi faccio abbindolare dal fatto che lei sia una dei 5 Stelle e quindi mi astengo o voto contro la sua posizione. Sarebbe assurdo, perché chi vota contro o si astiene è contro la Costituzione. Vorrei tanto far capire ai componenti del Gruppo MoVimento che non si può difendere la Costituzione e l'onestà se non attraverso l'applicazione dei principi della Costituzione. Credo non esista un esempio che calzi meglio all'articolo 68, che i Costituenti hanno voluto, affinché si verifichi la connessione con l'attività parlamentare. Sfido chiunque a dire che non vi sia connessione con l'attività parlamentare. Come leggete dalla proposta della Giunta, risulta che la senatrice in quest'Aula ha pronunciato determinate espressioni.

governare da odio e rancore verso una determinata persona *(Applausi)*, o avere soltanto un'interpretazione dei fatti preconcetta, basata su valutazioni soggettive.

Grazie

di parlare sull'ordine dei lavori. Il Gruppo Lega chiede la possibilità di sospendere per qualche minuto i nostri lavori per potersi riunire e consultarsi anche con le altre forze politiche sull'andamento di questa discussione. Senatore, non c'è una ragione evidente per la sua richiesta, ma cinque minuti di sospensione non si negano a nessuno.

Tra l'altro, devo dire con franchezza che non mi pare ci sia tutta questa differenza, a ben vedere e a leggere attentamente le dichiarazioni rese sia dal senatore Giarrusso che dalla senatrice Bottici, però sono fermamente convinto che anche in questo caso si tratti di applicare un principio e sono fermamente convinto che anche la vicenda della senatrice Bottici rientri nei casi di insindacabilità. Voglio ribadire per l'ultima volta

della Giunta delle immunità da ormai otto anni, e mi son sempre attenuto scrupolosamente all'osservanza delle leggi e della Costituzione. Quindi, il Gruppo di Italia Viva, come aveva fatto in Commissione, continuerà a ricercare l'osservanza della legge e della Costituzione e voterà a favore della proposta formulata dal relatore.

Senatore Pellegrini, la prego di prendere il suo posto. Senatore Castaldi, vada a sedersi al suo posto.

Ho una lunga esperienza, ma non ho mai visto per una insindacabilità tanta agitazione. È veramente inusuale. Quindi,

della proposta formulata dal relatore, sottolineando che continueremo ad osservare la legge e la Costituzione e rimarremo distanti dalle valutazioni di natura politica, così come sta accadendo, non solo in un organo paragiurisdizionale come la Giunta, ma è successo anche stamattina in un organo giurisdizionale, come il Consiglio di garanzia. Ho appreso infatti dai giornali che è stato violato il segreto della camera di consiglio di consiglio sulla decisione assunta ieri. Le decisioni dei giudici - perché tali sono i componenti del consiglio - non vanno mai discusse: sono quelle. Poi, ci sono gli strumenti che la legge appresta eventualmente per porvi rimedio qualora si ritengano sbagliate. continueremo - lo diciamo a voce alta - a osservare la Costituzione, che è il nostro credo, il faro che ci guida sempre nell'attività politica.

come si applica l'articolo 68 sull'insindacabilità, anche alla luce delle numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno valore di legge, si potrebbe citare esattamente questo caso. Infatti, in questo

che una certa *vis* polemica nasca da posizioni che possono politicamente esistere - e ci mancherebbe altro! - però, mi permetto di ricordare ancora, sperando di non essere pedante,

appartenenza, ma in sede di Giunta ci esprimiamo nel voto del singolo parlamentare, data la materia che riguarda le prerogative.

al Senato, non è più un qualcosa che appartiene al singolo; proprio perché stiamo parlando delle prerogative, appartiene all'Assemblea.

diciamo con un'assoluta tranquillità. Anche l'applicazione della legge è un elemento di garanzia per i cittadini, perché perché se non si condividono le leggi si possono cambiare, ma sussistendo, le stesse vanno applicate. Questo, però, vale anche per quelle considerazioni che a volte tendono a trasferire sul potere politico un'autonomia in base al fatto che si è ottenuto un consenso e un voto popolare. dovremmo tenere molto cari questi principi, indipendentemente dalle nostre idee, che possono essere diverse sulle singole questioni, perché il rispetto della legge è un principio di garanzia per tutti, salvo ovviamente quei casi previsti dalla Costituzione per cui, motivatamente, si possono avere diverse soluzioni. Gli unici casi

per manifestazioni di scontro, odio e rancore gli uni contro gli altri. Capisco che è difficile guardare con oggettività e indipendenza nel momento in cui sono sottoposti al nostro esame appartenenti a quest'Assemblea senatori che fanno parte di un Gruppo, però questo sforzo lo dobbiamo fare tutti perché l'articolo 68 della Costituzione è a garanzia dei singoli senatori, ma soprattutto della funzione che esercitiamo in questa sede. Pertanto, le appartenenze non dovrebbero

C'è una corrispondenza fra le dichiarazioni fatte in Senato e le dichiarazioni rese al di fuori. Non solo sono integralmente riportate, ma è detto e richiamato l'intervento fatto in Senato nel momento in cui si fa quell'intervista. Quindi, è una finalità divulgativa così evidente che non può far votare in maniera diversa, se non per l'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Bottici. Dichiaro, pertanto, il voto favorevole

pur rilevando che sul piano giuridico sussistono i requisiti rilevati dalla Corte costituzionale, rileva che sul piano politico si esprimerà contro la proposta, atteso che il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha sempre rinunciato all'immunità e ha sempre preferito sottoporsi al giudizio del magistrato come ogni cittadino». Ciò che ho appena letto non è ovviamente la dichiarazione di voto del mio Gruppo alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della senatrice Bottici, ma è un virgolettato estrapolato dal Resoconto sommario della seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, nella quale veniva esaminato proprio il caso della predetta senatrice. È chiaro che, decontestualizzato, non ci sarebbe nulla di male in quel virgolettato. È la semplice enunciazione di una linea che, giusta o sbagliata, potrebbe essere ritenuta legittima; tuttavia, non possiamo e non dobbiamo fingere di non sapere che, invece, qui un contesto c'è. Il contesto è serio e merita che si mantenga tale. Leggere nelle parole di un parlamentare del MoVimento 5 Stelle che il Gruppo MoVimento 5 Stelle avrebbe sempre rinunciato all'immunità sempre preferito sottoporsi al giudizio del magistrato come ogni cittadino - un'affermazione del resto ribadita poco fa da un appartenente al MoVimento - proprio mentre si sta esaminando la richiesta di autorizzazione a procedere di un parlamentare membro di quello stesso Gruppo, che si è appellato all'immunità concessa dall'articolo 68 della Costituzione, è un paradosso che non possiamo e non vogliamo accettare come senatori, ma ancora prima come cittadini italiani. La legge 20 giugno 2003, n. 140 non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. È chiaro, quindi, che se il caso in oggetto è arrivato all'esame della Giunta, prima, e dell'Assemblea, poi, è solo ed esclusivamente perché il parlamentare interessato dal provvedimento ha fatto ricorso alla prerogativa prevista dalla legge. Signor Presidente, personalmente accoglierei con favore la circostanza per cui il MoVimento 5 Stelle ha mutato radicalmente le proprie posizioni volte a rinunciare sempre e comunque ad avvalersi delle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione. Quello che invece continua a lasciarmi fortemente perplessa è constatare il comportamento altamente incoerente, visto che gli stessi, nel medesimo momento, da un lato utilizzano lo strumento e dall'altro si ostinano a negare le prerogative di cui all'articolo anche l'applauso va fatto stando seduti ai propri posti. che questa discussione non fosse così agitata perché non stiamo operando in una situazione di contrasto politico. Stiamo esercitando una funzione quasi giurisdizionale. Vi prego di ricordarlo e limitare

Per quanto mi compete, sono portata a ritenere che il tema di consentire ai parlamentari di svolgere il proprio compito con le garanzie e le tutele previste dalla legge sia ancor più importante e attuale oggi. L'avvento dei *social*, infatti, e l'uso troppo spesso incontrollato e irresponsabile degli stessi ci vede sovente, come politici, bersaglio facile per insulti e minacce per noi e i nostri familiari. A proposito di ciò, permettetemi di manifestare la mia assoluta vicinanza al segretario del mio partito, senatore Matteo Salvini, per i messaggi aberranti arrivati sui profili e che tutti noi abbiamo letto in questi ultimi giorni. Sono dispiaciuta di non aver visto, per il segretario Salvini, la solidarietà che avrei auspicato da più parti. Ne sono dispiaciuta, ma non totalmente stupita perché ho avuto modo a più riprese di sperimentare sulla mia pelle che, purtroppo, spesso gli stessi che a favore di telecamere si battono con ardore per l'abrogazione di privilegi di casta e per i diritti, all'ombra di un *post* non sono poi così solerti nello stigmatizzare comportamenti deplorevoli. È altresì doveroso rimarcare che tutte queste persone che oggi insultano sui *social* politici e non solo restano sempre - o quasi - impunite, come se fossero loro a godere di una forma inspiegabile di immunità. Nessuno chiede privilegi per i parlamentari; ciò che si chiede è solo il rispetto della legge, delle Istituzioni e della Costituzione. In conclusione, annuncio il voto favorevole alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. infatti convinti che sul piano giuridico sussistano i requisiti indicati dalla Costituzione e noi - almeno noi - quando siamo chiamati a esprimerci su casi di questo genere basiamo il nostro giudizio esclusivamente sullo studio dei documenti e sull'interpretazione della legge, a prescindere dal nome, dal partito e dalla storia del parlamentare in questione.

l'unanimità avrebbe dovuto contraddistinguere il voto in quest'Aula e anche perché credo ci sia una civiltà giuridica che dovrebbe orientare i nostri lavori. soprattutto quando si ragiona in termini giuridici, e io aggiungerei in verità anche politici, serve una linearità. All'interno della Giunta si è aperto un dibattito, che in verità non è ancora concluso del tutto, sul tema dell'interpretazione dell'articolo 68. L'articolo 68 è una prerogativa irrinunciabile da parte del parlamentare;

Questa prerogativa non può essere negata. Lo dico con molta tranquillità ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, perché l'errore che oggi fanno e che hanno fatto nei lavori della nostra Giunta è quello di saltare un articolo della Costituzione. la Costituzione non può essere applicata a pezzi e non si può bypassare un articolo perché non piace. Magari lo si cambia; ma un articolo della Costituzione va applicato. I lavori della Giunta consistono

questo ci porterebbe assolutamente fuori da un dibattito giuridico che deve essere a garanzia del lavoro e dell'importante ruolo che i parlamentari devono svolgere ora e domani per il Paese. Paese. Lo dico senza provocazioni: ho visto prima il collega Santangelo molto agitato, ma io ricordo che giustamente, a inizio legislatura, il collega Santangelo ha chiesto di essere audito dalla Giunta, ha portato le proprie ragioni e la Giunta ha accolto le ragioni del senatore Santangelo. Tutto questo ci porta ad avere una coerenza e una linearità. L'articolo 68, primo comma, non può essere bypassato. Noi non ci stiamo a cambiare opinione a seconda dell'evento o della persona coinvolta. Forza Italia voterà a favore della relazione del senatore Balboni, perché, al di là della veridicità delle affermazioni della senatrice Bottici al di là della loro gravità, è evidente che sono state svolte nell'esercizio del mandato parlamentare. Per questa ragione va salvaguardata non la senatrice Bottici, ma il mandato parlamentare come tale. Queste sono le ragioni per cui Forza Italia voterà a favore. Personalmente ritengo che anche la connessione tra l'attività *intra moenia* ed *extra moenia* del parlamentare vada rivista in maniera estensiva. Lo dico chiaramente ai colleghi, anche rispetto ad altre relazioni che ci interesseranno nel prosieguo della seduta. Abbiamo visto prima l'esempio del senatore Candiani, che addirittura era impossibilitato a svolgere un'attività parlamentare dal suo ruolo di Governo. Governo. Non si può ritenere che l'attività politica e parlamentare sia esclusivamente quella svolta in Aula. L'attività politica e parlamentare di un componente di questa Camera deve essere salvaguardata quando la si riconosce all'interno dell'attività politica e all'interno di un'attività tesa a garantire non solo

collega lamentarsi perché il senatore Gasparri non ha attribuito il ruolo di relatore a membri del MoVimento 5 Stelle.

oggi stiamo scrivendo possa servire a rafforzare la qualità e il lavoro di tutti i parlamentari, anche attraverso questa prerogativa irrinunciabile che Forza Italia difende oggi e difenderà sempre.

il caso specifico, pur rilevando che sul piano giuridico sussistono i presupposti rilevanti, ai sensi del dettato costituzionale, per la concessione dell'insindacabilità - in particolar modo per il nesso stringente che sussiste fra atto atto *extra moenia* e *intra moenia*, così com'è stato più volte riportato dai relatori - sul piano politico, però, non possiamo che esprimerci contro questa proposta della Giunta atteso che il MoVimento 5 Stelle ha sempre rinunciato all'immunità e ha sempre preferito sottoporsi al giudizio del magistrato, come ogni cittadino. *(Applausi)*. Questo è essere coerenti e non, come fa la Lega, che ci attacca, dice di essere contro e poi ripristina i vitalizi. Per questo, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, annuncio il voto contrario. Colleghi, vi invito a rimanere seduti e a smetterla con questa manifestazione. Non mi costringete a sospendere l'Aula,

mi costringete a sospendere la seduta. Procediamo con il voto. Cortesemente, riponete i vostri portafogli, mettetevi seduti e proseguiamo con i lavori d'Aula. Senatore De Vecchis, anche lei: che cosa facciamo, ci rispondiamo da uno scranno all'altro? Per cortesia.

ho sempre pensato che un politico si debba difendere nel processo e non dal processo. Lo pensavo prima di essere eletto e lo penso tuttora, tant'è che, quando sono stato querelato per diffamazione, non ho pensato neanche per un secondo di far valere l'insindacabilità di ciò che avevo detto. detto. Mi meraviglia, però, che è un esponente del MoVimento 5 Stelle non faccia altrettanto e non rinunci all'insindacabilità. Per questo motivo voterò contro il parere della Giunta che "scuda" la senatrice Bottici.

a questa prerogativa e al ruolo del Parlamento. Riesco però anche a capire le ragioni politiche del MoVimento 5 Stelle. Mi dispiace che da parte della senatrice Bottici non ci sia stata la rinuncia, che avrebbe forse tolto tutti dall'imbarazzo di questa discussione, mentre mi fa piacere avere assistito al passaggio molto moralista da parte del MoVimento 5 Stelle sul disgraziato ripristino dei vitalizi: peccato che arrivi da un Gruppo che ha confermato e conferma la fiducia di un amministratore delegato di una partecipata di Stato che è stato condannato per gravi reati finanziari, per avere falsificato i bilanci di Monte Paschi di Siena.

costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore,

nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) trasmessa dal Tribunale di Roma l'8 settembre 2020».

iscritto a seguito di querela proposta da tale dottoressa Rosanna Calzolari, magistrato presso il tribunale di sorveglianza di Milano, il 3 giugno 2020,

da precisare che il senatore Gasparri aveva anche chiarito che nel posto in cui lo stesso era stato mandato agli arresti domiciliari non vi era assolutamente alcun centro specializzato in problemi cardiologici.

Grazie La prerogativa dell'insindacabilità viene applicata a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, che è incentrato essenzialmente su due requisiti. Il primo, che è enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla corrispondenza di significato tra le opinioni espresse all'esterno e quelle espresse nelle aule parlamentari, Il secondo requisito per la configurabilità della prerogativa si basa sul cosiddetto legame temporale fra l'attività parlamentare e quella esterna.

A seguito anche di una discussione che, come sempre, è stata approfondita e si è incentrata proprio su questi temi di cui ho appena parlato, la Giunta aveva proposto a maggioranza di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri, che più volte ha ripreso questi temi anche nell'Aula del Senato, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e quindi ricadono nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta del relatore Cucca in ordine a questo procedimento penale che riguarda il senatore Maurizio Gasparri. Condivido pienamente le considerazioni di diritto svolte dal relatore: è dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la connessione tra l'attività parlamentare e le dichiarazioni *extra moenia* del senatore Gasparri. Mi permetto solo di aggiungere che, anche in questo caso, come in alcuni di quelli precedenti, non avrebbe dovuto esserci bisogno di arrivare

La critica politica riguarda l'attività di qualsiasi istituzione, compresa la magistratura. Non c'è un diritto della magistratura a non ricevere critiche, soprattutto quando si tratta di un magistrato che manda alla detenzione domiciliare un pericoloso criminale senza che ce ne siano i presupposti. *(Applausi)*. Da questo punto di vista, a maggior ragione, diamo convintamente il nostro voto favorevole alla proposta del relatore.

questo è un caso un po' diverso, perché non vi è dubbio che l'argomento in senso generale sia stato trattato in Aula, ma si

inserendomi in una discussione sollevata dal collega che mi ha preceduto, che ovviamente non è che non si possa criticare il rappresentante di un'altra istituzione (in questo caso stiamo parlando della giurisdizione), ma credo che, pur essendo l'argomento trattato sicuramente collegato, in questo caso vi sia un salto, perché si fa riferimento a una persona fisica individuata

il magistrato in questione dev'essere radiato dalla magistratura e il fatto che si chieda pubblicamente che il Consiglio superiore lo cacci su due piedi uno di quei casi in cui una valutazione non è superflua. Per questi motivi, come già fatto in Giunta, il nostro voto sarà di astensione.

ancora: «Cosa aspetta il CSM per radiarla dalla magistratura? Chiedo pubblicamente che il CSM la cacci su due piedi». Questa la frase nella sua completezza. Il problema è anche che questa frase, come viene rappresentato dalla querelante, ha scatenato sui *social media* più diffusi, quali Twitter e Facebook, tale dichiarazione, dandole ampia risonanza, scatenando un vero e proprio linciaggio mediatico. Ritengo però che il tema degli arresti domiciliari a detenuti ad alta pericolosità sia stato affrontato. Sono stato perfettamente d'accordo nel censurare

che, effettivamente, non è avvenuta. Da un punto di vista politico, quindi, il tema è stato molto diffuso e affrontato. Sebbene dalla relazione si desuma che l'interrogazione specifica è stata fatta in un tempo successivo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale fa intravedere la possibilità di una prevedibilità sul tema di un'interrogazione. Sotto questo profilo, quindi, il diritto di critica alle decisioni della magistratura non può essere certamente censurato. Il problema è quando poi si passa alla fase successiva, alla seconda affermazione, che riguarda la richiesta di provvedimenti disciplinari, che dovrebbero addirittura arrivare alla radiazione dalla magistratura di quel magistrato per l'esercizio di una funzione giurisdizionale (e quindi, tutto sommato, discrezionale), che può trovare anche mezzi di impugnazione o altri per sopperire alle eventuali deficienze del sistema o alla decisione non condivisa. Sotto questo profilo,

sia stata una sorta di eccesso nel diritto di critica, nel momento in cui si è richiesta questa radiazione, che ha provocato poi la gogna mediatica nei confronti del magistrato.

Signor Presidente, stiamo esaminando la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti del senatore Gasparri, nell'ambito di un procedimento penale che ha avuto origine da una querela presentata dalla dottoressa Rosanna Calzolari, magistrato presso il tribunale di sorveglianza di Milano, relativa a una dichiarazione rilasciata il 25 aprile 2020 dal senatore Gasparri a un'agenzia di stampa sull'operato della dottoressa stessa. Riguardo al lavoro del mio Gruppo, posso affermare con orgoglio che il nostro obiettivo, tanto in Giunta quanto in Aula, è stato sempre quello di assicurare tutte le garanzie costituzionali in tutti i casi in cui siano davvero in gioco i valori fondamentali della persona coinvolta, garantiti dal nostro quadro costituzionale e dalle carte internazionali. In particolare, in materia di insindacabilità, sottolineo che la nostra attività come Gruppo MoVimento 5 Stelle si è sempre basata su un'attenta disamina dell'attività del parlamentare indagato, in relazione alle tematiche per cui lo stesso viene querelato, considerando altresì che ogni situazione

ha solo espresso una critica politica legata alla questione delle scarcerazioni di pericolosi criminali a seguito dell'emergenza Covid. Rispondo che, se c'è stata una semplice critica politica, per di più avulsa dall'attività svolta dal parlamentare, ciò è ascrivibile a dinamiche di tutt'altra natura, che vanno risolte tramite le normali tutele ordinamentali, perché gli strumenti attualmente previsti per tutelare la libertà di espressione di ogni cittadino, che sia senatore o meno, ci sono e sono più che adeguate, tant'è che esprimere adeguate, tant'è che esprimere opinioni e critiche politiche oggi in Italia per fortuna non è assolutamente reato. Le frasi che il senatore Gasparri ha rivolto verso il magistrato sono ascrivibili a una critica estremamente aspra, per molti non accettabile, il relatore - che l'affermazione del senatore Gasparri sia chiaramente annoverabile al diritto di critica politica e, in quanto diritto, è in grado di escludere l'antigiuridicità della condotta. Mi chiedo pertanto perché il senatore Gasparri si appelli all'insindacabilità. Non è questa la sede per rilevare l'inesistenza del reato, che spetta invece alla magistratura ordinaria; non abbia quindi il senatore Gasparri di farsi giudicare, ma dimostri di avere fiducia nella magistratura. Teniamo anche ben presente che, ogni volta che ci si appella all'insindacabilità prevista della Costituzione, nello stesso tempo, si comprime gravemente il corrispondente diritto alla giustizia del cittadino querelante e questo è un gesto molto grave. Ecco perché l'insindacabilità può valere solo nei casi in cui si riscontra uno stretto nesso funzionale con l'attività parlamentare e non è allargabile a piacere, cioè non può essere applicata fuori dai casi previsti, mancando quindi i requisiti chiariti dalla giurisprudenza della Consulta, solo per il fatto di essere un parlamentare. *(Applausi)*. È una pretesa assurda e un'abitudine intollerabile, tipica di quell'odioso privilegio di chi si sente superiore ai normali cittadini.

e ancor più di un rappresentante dei cittadini in Parlamento come siamo noi. poi tutta una disamina molto attenta, però non voglio tediare l'Assemblea sul contenuto, che non collima con le affermazioni esterne; sul legame temporale, che non c'è; o sulla prevedibilità. posso dire tutte le date e tutti gli argomenti di cui parlava, come le carceri che hanno bisogno di più pene alternative per evitare problemi di malattie, invece adesso per quella esterna critica l'applicazione delle pene alternative; insomma, andiamo avanti. assolutamente macroscopico e oggettivo, mancano completamente i requisiti necessari per concedere l'insindacabilità richiesta, eppure si vuole sfruttare comunque il privilegio. Questo è profondamente sbagliato, ma il problema è anche un altro: occorre fare grande attenzione ai messaggi d'odio che si lanciano, perché potrebbero generare un effetto domino emulativo, come ha già evidenziato il collega Grasso, quello che la stessa querelante definisce un vero e proprio linciaggio mediatico. Facciamo quindi attenzione ai messaggi d'odio. Termino il mio intervento, dicendo che per questo caso spetta alla magistratura la valutazione e ribadendo che ignorare i limiti tracciati della Corte costituzionale è suscettibile di svilire la prerogativa in questione, trasformandola in un privilegio personale e quindi in una sorta di impunità del tutto inaccettabile. Per questi motivi, annuncio che il MoVimento 5 Stelle voterà in modo contrario rispetto alla proposta di insindacabilità formulata dal relatore. simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione).* Senatore Candiani, non ritiene che bisognerebbe stare in Aula quando indìco la votazione?

68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) trasmessa dal Tribunale di Trapani il 17 novembre 2020». elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo

la relazione che ho già depositato, per far presente all'Assemblea che si tratta di una querela depositata dal signor Biagio Bosco nei confronti del senatore Giarrusso per alcuni commenti pubblicati su Facebook. In particolare, la frase incriminata sarebbe la «Caspita! Persino i mafiosi intervengono adesso! Siamo proprio alla mafia 2.0». In relazione a questa frase incriminata, il senatore Giarrusso ha chiarito in modo molto preciso che esisteva una corrispondente attività parlamentare *intra moenia* che giustificava tale affermazione. Mi richiamo alla mia relazione, perché è ben chiarito come il senatore Giarrusso si sia a più riprese occupato del tema della mafia, in particolare nella provincia di Trapani. Come se non bastasse - questo per me va sottolineato e chiedo all'Assemblea di ascoltarmi con un attimo di pazienza - siamo di fronte a una strana fattispecie: la querela è presentata dal signor Biagio Bosco; tuttavia, analizzando tutti i *post* che sono stati pubblicati sulla pagina Facebook, ci rendiamo conto che la frase incriminata è stata pubblicata prima

Ancora una volta, siamo di fronte a un magistrato che trova più comodo mandare a noi gli atti anziché leggerli con la dovuta attenzione, motivo per cui, a maggior ragione, propongo all'Assemblea

e l'oggetto della condotta presa in esame si riferisce ad altra persona. Mi sembra quindi molto pacifico ed evidente che non può che esserci un voto favorevole alla proposta del relatore Balboni.

le motivazioni addotte nella relazione del senatore Balboni, atteso che non c'è assolutamente coincidenza tra il destinatario della dichiarazione del senatore Giarrusso, che è riferibile come commento al signor Ugo Gaspare Lazzara, e il querelante, che è invece il signor Bosco. Mancano quindi mancano proprio i presupposti per qualsiasi valutazione sull'insindacabilità.

Signor Presidente, nonostante, come già detto, dai documenti depositati in Commissione si evidenzi la possibilità che non vi sia una corrispondenza tra querelante e soggetto destinatario della dichiarazione del senatore Giarrusso, preannuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle rispetto alla proposta conclusiva della Giunta, rilevando che nel caso di specie l'unica autorità legittimata a valutare la sussistenza o meno del reato di diffamazione è la magistratura. L'insindacabilità non può costituire il pretesto per configurare un indebito privilegio a beneficio dei soli parlamentari. pertanto che in questo caso non ci sarà alcun tipo di problema per il soggetto querelato nel dimostrare l'infondatezza della querela dinanzi al giudice ordinario. proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo

elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso una procedura di mediazione civile presso l'Organismo di mediazione forense di Roma nei confronti della senatrice Anna Maria Bernini, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

Si tratta solo di evidenziare un fatto: nella fattispecie - e ciò è stato oggetto di una certa discussione in Giunta - la vicenda civile era ancora nelle fasi preliminari davanti all'organismo di mediazione. Poiché ancora non c'era un procedimento, ci si era posti il problema se effettivamente si potesse intervenire o meno. Tuttavia, laddove la mediazione sia

in questo senso, si è deciso di esprimere parere favorevole all'insindacabilità delle opinioni espresse. Voglio ricordare che, come leggerete nella relazione depositata e distribuita,

in un'infinità di circostanze, fin dalla scorsa legislatura, aveva già espresso, ha detto: «un accanimento mai visto né a livello nazionale né internazionale; è l'unico processo che riesce ad andare a buon fine perché tutti gli altri sono finiti miseramente; (...) non è una eccentricità, questa è una violazione di tutti i precetti democratici costituzionali...», annunciando anche la richiesta di una Commissione di inchiesta sull'intera vicenda. è innegabile che la senatrice Bernini a più riprese abbia pronunciato esattamente le medesime parole sia espressa con i medesimi termini. È pertanto evidente che sussistono i requisiti previsti dalla Costituzione per il riconoscimento dell'insindacabilità e, in questo senso, la Giunta ha deciso a maggioranza di riconoscere

Signor Presidente, vorrei leggere all'Assemblea le frasi pronunciate dalla senatrice Bernini

Queste le frasi pronunciate dalla senatrice Bernini in relazione alla condanna inflitta all'onorevole Berlusconi, di cui tutti siamo a conoscenza: «Un accanimento «Un accanimento mai visto né a livello nazionale né internazionale»; «questo è l'unico processo che riesce ad andare a buon fine perché tutti gli altri sono finiti miseramente»; «Però - lo ripeto - questa non è una eccentricità, questa è una violazione di tutti i precetti democratici costituzionali... se viene meno la terzietà del giudice, lei capisce è una cosa terribile il venir meno dell'indipendenza del giudice, significa la totale perdita della credibilità della magistratura». «Una Commissione d'inchiesta che finalmente faccia chiarezza proprio su quello che voi state raccontando, cioè su questi intrecci, questi nodi gordiani tra politica e giustizia»; «lo sconcio più enorme dopo la sentenza del 2013 è quella del 27.11.2013 27.11.2013 quando in Senato Berlusconi è stato scacciato in maniera indecente, illegittima, indegna, sulla base di una sentenza che ora si dimostra totalmente infondata... perché quello che la sinistra non è riuscita a fare per ventiquattro anni, cioè, battere Berlusconi, lo si è fatto per mano magistratuale, questa è la vergogna, questo è lo sconcio, che noi dobbiamo raccontare

Questa è la frase che la senatrice Bernini stava commentando. Guarda caso, proprio due giorni fa, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rivolto all'Italia dieci domande per capire se il processo a Berlusconi rispettava le regole di equità, di giustizia e di contraddittorio. Allora in quest'Aula non solo dico che non solo voterò a favore della proposta del relatore, ma mi assumo ogni responsabilità nell'affermare che quei due magistrati si devono vergognare e non meritano

Signor Presidente, direi che con questo caso possiamo proseguire il nostro confronto

seppure capisco che è quasi un'occasione imperdibile. Tuttavia, voglio ribadire che è un classico caso in cui una collega in una

Ovviamente difendo il diritto della senatrice Bernini a esprimere pienamente le proprie posizioni,

le capacità e le sedi per confrontarsi esattamente sul merito delle dichiarazioni della collega. Dichiaro quindi il voto favorevole sulla relazione.

che all'articolo 3, comma 2, richiede che ci sia un procedimento giurisdizionale pendente e sia eccepita dall'interessato l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione; a seguito dell'eccezione, il giudice dispone l'invio degli atti alla Camera a cui il parlamentare appartiene. L'articolo 3, comma 7, della citata legge prevede anche che la questione dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione possa essere posta direttamente dal parlamentare. Tuttavia, anche in tale caso deve essere certamente in corso il procedimento giurisdizionale, come la stessa norma

Proprio per questa motivazione, ritengo che ci si debba astenere dal giudizio e, quindi, attendere eventualmente l'inizio di un procedimento giurisdizionale per poter affrontare la questione nel merito.

intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Lega alla proposta presentata. La controversia in atto ha ad oggetto dichiarazioni rese dal dottor Nicola Porro, dal dottor Sallusti, dal dottor Sansonetti e dall'onorevole

che hanno fatto parte della sezione feriale che ha pronunciato una sentenza nel 2013 assunta nell'ambito della vicenda giudiziaria nota come vicenda Mediaset nelle cronache giornalistiche. Con la predetta sentenza è stato rigettato il ricorso, tra le altre statuizioni, del senatore Berlusconi avverso sentenza di Corte d'appello di Milano del 2013. Secondo i dottori Esposito e D'Isa, nel corso delle puntate del predetto programma televisivo, il conduttore Porro e i suoi ospiti avrebbero operato una ricostruzione distorta e ingannevole dei fatti relativi alla citata vicenda, con commenti fuorvianti. Nel corso della puntata del 13 luglio 2020 veniva invitata anche la senatrice Anna Maria Bernini. All'inizio della trasmissione, annunciata dal titolo «Nuovo documento sulla sentenza Berlusconi», il conduttore Porro riportava, ad avviso degli istanti, in maniera sintetica, generica e non conforme al contenuto, le contestazioni sollevate da questi ultimi e la richiesta di rettifica del 30 giugno 2020 inerente alle affermazioni del defunto giudice Amedeo Franco. Successivamente il dottor Porro riportava la notizia della denuncia avanzata dal dottor Esposito nei confronti di tre dipendenti dell'albergo di Ischia che avevano attribuito a quest'ultimo gravi affermazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, mandando nuovamente in onda le dichiarazioni degli interessati. Riferiscono gli astanti che la senatrice Bernini pronunciava, a tal proposito, i seguenti commenti: «un accanimento mai visto a livello nazionale, né internazionale»; «questo è l'unico processo che riesce ad andare a buon fine perché tutti gli altri sono finiti miseramente». È evidente la legittimità di tali affermazioni, che costituiscono un palese esercizio del diritto di critica politica da salvaguardare e tutelare. Un consistente ambito dell'attività parlamentare della senatrice Bernini è riferito all'esercizio della giurisdizione nel nostro Paese. Numerosi Numerosi sono gli interventi che si sono susseguiti in Aula e gli atti parlamentari che la relazione della Giunta individua nel dettaglio. Il 27 novembre 2013 si registra un intervento della senatrice in Aula a favore della convalida del senatore Berlusconi, durante il dibattito sulla proposta di decadenza in applicazione della cosiddetta legge Severino. In tale occasione, la senatrice ha ribadito più volte l'accanimento nei confronti del senatore Berlusconi, pronunciando le seguenti frasi: «Oggi siamo chiamati a stabilire se il Parlamento [...] abdica alla sua funzione, limitandosi a scrivere la pagina definitiva di un uso politico della giustizia che dura da vent'anni». Una settimana prima della trasmissione televisiva, il 6 luglio 2020, il Gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato ha presentato un disegno di legge, di cui la senatrice Bernini è prima firmataria, avente ad oggetto l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale sull'uso politico della giustizia, recante il numero 1870. L'articolo 1 del disegno di legge elenca gli obiettivi di tale Commissione, tra i quali in particolare si evidenziano l'influenza diretta o indiretta delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sui comportamenti dell'autorità giudiziaria, sia inquirente che giudicante, ma anche se e in quale misura singoli esponenti o gruppi all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio democratico e con il principio di sovranità popolare, in particolar modo diretta a interferire con attività parlamentari e di Governo e, più in generale, con l'esercizio delle funzioni di altri organi costituzionali. Nella relazione del predetto disegno di legge si legge testualmente: «In questo vuoto del sistema politico, si è inserita la magistratura, quella al suo interno fortemente politicizzata, almeno negli organismi di vertice». Queste sono alcune dichiarazioni *intra moenia* significative, che sono idonee a radicare la prerogativa dell'insindacabilità, nel caso di specie ancora più pregnante essendo volta a garantire il diritto di critica del parlamentare rispetto al potere giudiziario, diritto che in tal caso deve assumere una valenza rafforzata, atteso che, se al parlamentare fosse preclusa la facoltà di esprimere le proprie valutazioni politiche rispetto alla magistratura e ai magistrati, tale limitazione sarebbe suscettibile di attenuare il ruolo del Parlamento e la sua autonomia rispetto al potere giudiziario, che è innanzitutto autonomia di critica e di giudizio. Signor Presidente, in questo intervento vorrei essere ancora più breve, giacché ho già detto tanto nei precedenti interventi. Mi vorrei limitare soltanto a dire, in merito al caso della senatrice Bernini, di lasciar stare la ricerca spasmodica di requisiti giustificativi, scartabellando nei vari atti per cercare la frase a cui radicare il nesso funzionale. Invece di cercare nessi troppo generici, legami temporali che sono troppo labili o arrampicarsi e sforzarsi per trovare il legame nella plausibile prevedibilità o non prevedibilità di un atto successivo, io chiedo alla senatrice Bernini, che non mi sembra una persona timida, che sa argomentare (glielo riconosco) e che saprebbe ben difendersi in un'aula di tribunale, se non sarebbe stato più opportuno per lei affrontare la situazione direttamente.

non è questo lo spirito della norma; è ben altro. Chiediamoci invece se sono in gioco i principi dello Stato democratico: non credo. Chiediamoci se si tratta di pericolose spallate del potere giudiziario per demolire il potere legislativo oppure no, se sono questioni molto meno gravi. Qui non c'è nemmeno un vero processo; si parla di udienze di mediazione, che spesso si chiudono lì, senza andare a processo. Quindi brevemente io dico: si vuole concedere l'insindacabilità? Facciamolo; ma facciamolo solo in casi alti, eccezionali, importanti (non in questo), così da rispettare il progetto originario dei nostri Padri costituenti. Non svilite questo importante istituto *(Applausi)*, che avete ridotto a un'inaccettabile impunità o, peggio ancora, a un privilegio odioso, tipico di chi crede di essere superiore ai normali cittadini. Allora, colleghi, facciamo la cosa giusta e per fare la cosa giusta e per i motivi descritti

simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto, per il quale è in corso una procedura di mediazione civile presso l'Organismo di mediazione forense di Roma nei confronti della senatrice Anna concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione).*

Ora, la linea si stava peggio quando si stava peggio è inaccettabile perché il signore che lamenta il fatto che quando c'erano i chioschi le spiagge erano ben tenute dimentica di dire che quei chioschi erano illegali e governati dalla mafia». La richiesta ovviamente è riferita all'ultima parte delle affermazioni del senatore Mirabelli, ma è assolutamente in linea con quanto da lui stesso sempre affermato nell'ambito della sua attività in Commissione

dopo che la domanda era stata proposta all'organismo di mediazione e avevamo radicato il procedimento, sono stati poi notificati, ed è stato difficilissimo recuperarli, anche gli atti di citazione. La vicenda è estremamente chiara se solo si considera che in tutte le affermazioni del senatore Mirabelli, comprese quelle rilasciate nel corso della trasmissione, il senatore non ha fatto alcun riferimento specifico e personale a nessuno, neanche a quelli che poi lo hanno citato in giudizio. Ha semplicemente parlato genericamente della vicenda dei chioschi sul litorale di Ostia,

La relazione della senatrice Modena è ben motivata e il nesso funzionale è fuori discussione.

chi non ne fa parte, oggi ha partecipato ad una giornata di approfondimento e di discussione. proprio l'applicazione della funzione del parlamentare che, tra l'altro, facendo parte della Commissione antimafia, esercita il ruolo di indagine sotto il profilo politico di fenomeni talmente gravi che hanno motivato la costituzione di una Commissione *ad hoc* ed esercita questo ruolo come deve esercitarlo, riportando pubblicamente non solo i punti e gli esiti, ma denunciando politicamente un fenomeno ed esercitando il ruolo politico sul piano della

pieno dell'attività del parlamentare e di tutela delle sue libertà nei confronti di altri tipi di pressioni, esattamente lo spirito con cui è stato scritto l'articolo 68 della dichiaro il voto favorevole in relazione alla prospettazione che è stata fatta perché è evidente in questo caso che il senatore Mirabelli non ha fatto che rappresentare ciò che era emerso chiaramente nel corso della XVII legislatura in Commissione antimafia relativamente alle problematiche del litorale di Ostia in particolare, sulle otto spiagge libere, sui chioschi su cui doveva decidere l'amministrazione comunale circa la gestione, sul clima di vero e proprio *racket* di intimidazione che operava in quel litorale. Le sue dichiarazioni coraggiose, quindi, non hanno certamente tradito il divieto di divulgazione di qualcosa che era già

senza indicare soggetti, senza indicare particolari tali da consentire di individuare delle persone offese. La querela è stata presentata da persone che si sono autoqualificate come

della Giunta che ha dichiarato l'insindacabilità delle dichiarazioni espresse dal senatore Mirabelli. Per ragioni di logica, ma anche di tempo, mi riporto alla relazione che condividiamo *in toto* esposta poc'anzi dalla relatrice Modena. Voglio dare atto anch'io, durante questo mio breve intervento, dell'attenzione e del coraggio del senatore Mirabelli nel fare

hanno fatto propri degli indirizzi della Corte europea dei diritti dell'uomo, dimostrando che c'è una connessione tra le dichiarazioni *extra moenia* del senatore, rilasciate nel caso di specie in televisione, e il lavoro che ha svolto da parlamentare *intra moenia*, ovvero all'interno delle istituzioni. Diversi sono i casi nei quali è stata certificata

al 2016, quindi gli consiglio di non stare a cercare ancora requisiti nei vari discorsi vecchi di anni, a ritagliare una frase a cui radicare il nesso funzionale, a sforzarsi di trovarsi per fortuna o per caso dentro il legame temporale. PRESIDENTE. Senatrice, deve rivolgersi alla Presidenza, non è un dibattito fra lei e il senatore Mirabelli.

guardando il mio foglio. È un uomo leale, retto, di spessore morale, glielo riconosco io ma glielo riconoscono tantissimi colleghi. È un uomo che non cede certo alle intimidazioni dei chioschi del litorale laziale. Ma io mi chiedo se non sia più dignitoso e corretto per lui presentarsi in giudizio e far dichiarare l'inesistenza del reato, perché il reato non c'è, ci mancherebbe, massima solidarietà per il senatore Mirabelli. Facciamo però uno sforzo di coraggio e di dignità, diamo alla prerogativa dell'insindacabilità il valore che merita, quello di strumento importante che previene e contrasta la prevaricazione dei poteri dello Stato per preservare proprio l'equilibrio della forma democratica. Concediamola solo in casi gravi, eccezionali e importanti, così da rispettare il sogno e il disegno dei padri costituenti. Siamo sempre allo stesso punto. Non sviliamo questa prerogativa fino a farla inevitabilmente assomigliare a un privilegio della classe politica. Questo va assolutamente evitato! In conclusione, per tutti questi motivi, non ritengo opportuno concedere l'immunità e, valutando che questo caso vada risolto dalla magistratura ordinaria, annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

non ho condiviso le sue posizioni, ma ho apprezzato la sua serietà e il suo impegno, all'interno soprattutto della Commissione antimafia. L'ultimo intervento mi ha scioccato. Nei casi precedenti si poteva anche fare una valutazione politica, discutibile o no, ma in questo caso, nel quale in maniera eclatante il collega Mirabelli, assumendosi la propria responsabilità e sottraendosi al timore di ritorsioni, ha denunciato fatti che poi successivamente sono stati dimostrati come reali, annunciare un voto contrario, significa stracciare la Costituzione! Significa abolire la Costituzione! Significa tornare all'età della pietra! Significa imbarbarire il Parlamento! E di questo dovete solo vergognarvi!

presso l'Organismo di mediazione forense di Roma, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione).*

«Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 16519/2017 RGNR - n. 8701/2017 RG GIP) trasmessa dal Tribunale di Napoli-Nord Sezione del Giudice per le indagini preliminari il 13 aprile 2018».

di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria per le telefonate del 20, 22, 23 marzo 2015, 1° aprile 2015 e 5 maggio 2015 e di respingere invece la stessa limitatamente alla telefonata del 10 aprile 2015; per quel che concerne le conversazioni intercettate sull'utenza telefonica di Angelo Liccardo, di accogliere l'istanza del giudice per le indagini preliminari limitatamente alla telefonata del 16 marzo 2015 e di respingerla invece per la telefonata del 14 aprile 2015. Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

alla Giunta, quindi abbiamo provveduto ad esaminarla. in maniera molto chiara e precisa nella relazione depositata. Voglio solo precisare che anche in questa circostanza, come in tutte le altre delle quali la Giunta si è occupata nella materia dell'utilizzo delle intercettazioni, abbiamo applicato il consueto principio - è ben spiegato nella relazione e, quindi, evito di riproporlo in questa sede per non allungare troppo i tempi - di dichiarare l'utilizzabilità esclusivamente delle intercettazioni che sono sicuramente casuali,

che uno dei due interlocutori fosse un parlamentare. Nella fattispecie questo lo si può desumere agevolmente perché la prima è una telefonata che casualmente fa una persona sottoposta a intercettazioni telefoniche, e una a intercettazioni telefoniche, e una persona che parla con il soggetto intercettato viene ascoltata per la prima volta: è verosimile quindi - ed è questo il principio che è sempre stato applicato in questa materia e che abbiamo fatto nostro in Giunta nostro in Giunta - che chi ascoltava non poteva certamente sapere, durante quella prima intercettazione, che l'interlocutore del soggetto intercettato fosse un parlamentare. Seguendo Seguendo questo profilo logico, si suppone che siano ancora casuali quelle intercettazioni che si sono susseguite a distanza di un brevissimo lasso di tempo. È ancora verosimile, conoscendo come funziona il sistema delle intercettazioni, che in una o due giornate, quando cioè vengono solo compilati i brogliacci, ma non sono ancora esaminati nel merito e soprattutto non si è ancora verificata quale sia quale sia l'identità del soggetto che dialoga con il soggetto intercettato, si considerino casuali soltanto quelle. In questo senso trova motivazione la decisione, assunta

non sia venuta a conoscenza che l'interlocutore fosse un parlamentare. Lo stesso criterio è stato applicato anche per le intercettazioni sull'utenza di tale Liccardo e, quindi, si è

conosceva l'identità dell'interlocutore o, in caso negativo, avrebbe potuto certamente conoscerla. Questo è il senso con cui si è preso la decisione a maggioranza ed è questa la proposta che la Giunta formula all'Assemblea.

intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta del relatore, che tra l'altro ho votato

ben spiega il senatore Cucca nella sua relazione, ed è ciò che ci consente di entrare nel merito. Riteniamo quindi giusto autorizzare l'utilizzo di tutte quelle telefonate che rivestono

e di captare conversazioni riguardanti un parlamentare. Le uniche due intercettazioni sulle quali la Giunta nega l'autorizzazione sono molto avanti nel tempo, per cui non è plausibile immaginare che gli inquirenti non fossero in realtà già a conoscenza, per il tempo trascorso, Grazie

Grazie Signor Presidente, colleghi, anche in questo caso il nostro voto sarà favorevole. Mi preme sottolineare che il documento è arrivato al nostro esame già con una prima selezione fatta dal giudice per le indagini preliminari nel ruolo che gli è proprio, e cioè quello di essere lui innanzitutto a giudicare se possa essere accolta la richiesta del pubblico ministero. Questo avviene per le intercettazioni, le richieste di arresto e quant'altro; nel caso in esame il giudice per le indagini preliminari ha già escluso dalle richieste fatte al pubblico ministero l'utilizzabilità di alcune conversazioni, in quanto, trattandosi di utenze dei familiari,

perché è evidente che noi non facciamo un processo parallelo, ma valutiamo le argomentazioni a sostegno della richiesta. Quindi, abbiamo valutato la rilevanza e l'indispensabilità

quando è chiaro che l'obiettivo non può che essere quello del parlamentare per il punto e la situazione in cui si trovano le indagini. Quindi, abbiamo ritenuto di autorizzare

Annunciamo il voto favorevole sulla deliberazione della Giunta. Coerentemente con quanto già deliberato, usata per riconoscere la casualità delle intercettazioni e, quindi, la necessità di verificare, solamente in relazione a questa, la possibilità di autorizzazione

hanno la caratteristica di casualità, determinante anche dal fatto che, per la loro vicinanza, gli inquirenti non avevano certamente contezza del fatto che il terzo indagato interloquisse con un parlamentare coinvolto in vicende di rilievo penale, così pure per quanto riguarda la telefonata del 10 aprile 2015. 2015. Siamo d'accordo che vada accolta l'istanza sull'utenza telefonica del Liccardo per la telefonata del 16 marzo 2015, mentre va respinta per la telefonata del 14 aprile 2015. È infatti plausibile che sia avvenuto un mutamento della direzione dell'atto di indagine rivolta verso il parlamentare. Annuncio pertanto il voto favorevole alla richiesta della

annuncia il voto favorevole alla relazione del senatore Cucca, che ci ha trovato d'accordo sulla concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni delle conversazioni del 20, 22 e 23 marzo,

infatti, che in questo caso andavano rigorosamente applicate la legge e la sentenza della Corte costituzionale, la n. 390 del 2007.

possono essere utilizzate solo se occasionali, fortuite; quindi, non deve essere trascorso un notevole lasso di tempo, lasso di tempo, il quale consente alla magistratura di sapere che sta intercettando un parlamentare per cui è obbligata a chiedere preventivamente l'autorizzazione alla Camera di appartenenza. Quindi, anche in questo caso si deve escludere per quelle intercettazioni il *fumus persecutionis*

era chiaro alla magistratura che stava captando un parlamentare, per cui è sopravvenuto il mutamento di direzione dell'atto di indagine. Per questi motivi confermo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

di alcune intercettazioni; non sono d'accordo sulla parte che denega la possibilità per le restanti. Ho chiesto in Giunta di poter votare per parti separate e questo non è stato consentito.

perché nella parte in cui le intercettazioni vengono denegate si sostiene che le stesse siano state captate senza che ci fosse casualità. In realtà, sia per la distanza temporale delle stesse intercettazioni l'una dall'altra sia perché, comunque, gli intercettati erano tutte persone indagate, che sono state captate in momenti del tutto casuali in conversazioni con il senatore Cesaro, sarebbe stato molto più corretto poter votare per parti separate.

per quel che concerne le conversazioni intercettate sull'utenza telefonica di Antonio Di Guida, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria per le telefonate del 20, 22, 23 marzo 2015, 1° aprile 2015 e 5 maggio 2015 e di respingere invece la stessa limitatamente alla telefonata del 10 aprile 2015; per quel che concerne le conversazioni intercettate sull'utenza telefonica di Angelo Liccardo, di accogliere l'istanza del Giudice per le indagini preliminari limitatamente alla telefonata del 16 marzo 2015 e di respingerla invece per la telefonata del 14 aprile 2015. *(Segue la votazione)*.

Grazie

elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria. Chiedo al relatore, senatore Durnwalder, se intende intervenire. Signor Presidente, abbiamo in esame la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti dinanzi al tribunale di Bologna per concorso nei reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio

primo comma, del codice penale e nonché per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, aggravati ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del codice penale. Come già ricordato dalla Presidente, la Giunta nella seduta del 1° luglio 2020 ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata, ossia quella del 30 marzo 2013, e di respingerla per le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, del 27 giugno e del 10 luglio. Per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, propone di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria con riguardo alla prima telefonata, ossia per quella del 30 marzo 2013, per la quale è stata riconosciuta l'occasionalità della medesima. Le telefonate, invece, dell'8 giugno, del 27 giugno e del 10 luglio 2013 sono state effettuate diverso tempo dopo la prima telefonata del 30 marzo 2013. Tale elemento costituisce un sintomo del mutamento di direzione dell'atto di indagine, apparendo implausibile che l'autorità giudiziaria non si sia accorta del coinvolgimento di un parlamentare dopo tanto tempo. L'utilizzo dei tabulati richiede, invece, la verifica se ci sia o no un *fumus persecutionis*. Non c'è il *fumus* di primo grado, atteso che nessun elemento rende verosimile un'inimicizia o, comunque, un intento persecutorio perseguito dal magistrato. Parimenti non è configurabile un *fumus* di terzo grado consistente nel carattere manifestamente infondato degli atti in questione, atteso che non è emerso alcun elemento tale da ritenere *ictu oculi* evidente una supposta incongruità o una supposta palese illegittimità degli atti.

Signor Presidente, la questione in oggetto va avanti da molto tempo e si riferisce al ruolo che Carlo Giovanardi, all'epoca in cui era senatore, ha svolto in sede delle procedure relative alla ricostruzione dopo gli eventi sismici che hanno colpito l'area interessata. A Giovanardi A Giovanardi è stato ascritto di aver commesso dei reati, per i quali è indagato, avendo perorato delle cause di aziende escluse dalla cosiddetta w*hite list* - probabilmente si usa un termine straniero perché un concetto del genere

persone legate alla criminalità organizzata). Un caso emblematico e non unico

Sta di fatto che il senatore Giovanardi si adoperò perché questa preclusione all'inserimento nella w*hite list* Non è mai stato neppure ipotizzato che il senatore Giovanardi abbia ricevuto, in cambio di questa presuntamente illecita attività, qualsiasi tipo di

virulenza la propria posizione e di aver pronunciato delle frasi che sono poi state indicate come reato (a livello di minacce e così via). si debba prestare una particolare attenzione su un argomento di questo genere. Se un parlamentare si batte contro una vicenda che a lui pare una palese ingiustizia, senza alcun tipo di convenienza che non sia quella di perseguire la giustizia per un'azienda del territorio che l'ha eletto e che in ogni caso egli rappresenta (ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione),

possiamo ritenerci tutti coinvolti - che il mandato parlamentare consista non soltanto nel venire qui a premere qualche bottone su indicazione altrui,

Mirabelli, la vasta maggioranza del Senato ha giustamente ritenuto esercitare la sua funzione di parlamentare nell'aver formulato accuse a certi ambienti che poi la magistratura stessa ha ha indagato e ha riconosciuto come legati alla criminalità. Qui abbiamo un caso simile: un senatore si adopera per evitare un'ingiustizia e per questo viene intercettato, contro i principi della Costituzione. Ricordiamo che non c'è solo l'articolo 68 della Costituzione, ma c'è anche l'articolo 15, che protegge la riservatezza nelle comunicazioni tra tutti i cittadini. Il parlamentare ne ha un'altra in più,

evitare il rischio che una parte possa sapere cosa sta facendo, a cosa sta lavorando e come si sta organizzando l'altra parte. Questo non è ammissibile. Se poi ciò avviene prendendo a pretesto il fatto che uno si batte per difendere la giustizia, per difendere le esigenze del territorio o per difendere dei posti di lavoro, ebbene, questo diventa particolarmente preoccupante.

l'Assemblea, come ha ricordato poco fa il senatore Malan. La vicenda che ha investito il nostro ex collega Giovanardi, che è stata oggetto anche di dibattito in Giunta e su cui il relatore Durnwalder

alla natura e alla sostanza dell'articolo 68 della Costituzione e dell'attività parlamentare. Oggi in molti interventi - lo ho fatto anche il presidente Grasso - si è discusso della contestualità e se l'interrogazione su un determinato fatto sia arrivata in un tempo congruo, profilo di cui anche

e successivamente prende non dico più carta e penna, ma l'iPad o l'iPhone, e scrive l'interrogazione. Gli stessi Uffici del Senato sono spesso molto attenti - e questo è doveroso - quando le interrogazioni investono i rapporti tra magistratura e politica.

da interlocutori che registravano la telefonata. Poi quelle registrazioni, che non sono intercettazioni, vanno in mano alla magistratura, che non sappiamo ancora se le utilizzerà o no. C'è stata una corrispondenza a questo scopo tra la Giunta, che ha condiviso all'unanimità la richiesta di informazioni, e la Presidenza del Senato, perché è la Presidenza del Senato che scrive al tribunale. È quindi una vicenda in cui alcuni interlocutori e vedo il senatore Durnwalder che, in qualità di relatore

La vicenda Giovanardi, che è un caso concreto, e non una vicenda di riflessione politica, che avrà sviluppi ulteriori quando torneremo in Assemblea con le registrazioni fatte da un signore, porta ad affermare che almeno le intercettazioni devono essere autorizzate, decise dalla magistratura e, nel caso di un parlamentare, se non sono casuali e si ripetono, bisogna chiedere l'autorizzazione. Invece l'interlocutore di Giovanardi ha registrato il colloquio e lo ha dato alla magistratura. In una conversazione privata io posso dire che mi sta antipatico il senatore Mirabelli o altre cose. Se però penso che sia una conversazione privata, è complicato poi configurare un reato. Se tutte le conversazioni private che facciamo

parlamentari - anche con la foga che gli è propria. Qualcuno ha conosciuto Giovanardi e si è imbattuto nel suo modo, a volte anche impetuoso. Ricordo che una volta ha detto che andava in prefettura e sparava a tutti. Lo ha detto però come uno che parla a dei tifosi: nessuno può immaginare Giovanardi entrare in prefettura a mano armate fare una strage. Anche su questo c'è un'indagine in corso per non so quale reato avrebbe compiuto in strada, parlando con delle persone. Quindi si possono censurare il linguaggio e il comportamento. Sulla vicenda

condannati; alcuni magistrati sono stati trasferiti nell'ambito delle polemiche e delle discussioni che si sono dipanate dopo la vicenda Palamara.

collega. Ci sono colleghi anche in questa legislatura che hanno firmato delle interrogazioni parlamentari; se uno vuol fare una congiura, non fa certamente interrogazioni parlamentari, interventi in Assemblea o va in prefettura sostenendo con vigore le proprie ragioni. Non credo che uno che voglia fare una congiura agisca utilizzando la propria condizione di parlamentare. Ecco perché le vicende di Giovanardi vanno sulla sostanza dell'articolo 68 della Costituzione. Anche i colleghi che contestano l'articolo 68 dalle

vicenda di cui stiamo discutendo, per la delicatezza di questo episodio e di quelli che seguiranno, c'è da fare una riflessione, che abbiamo fatto con delle discussioni apposite che riguarda il Parlamento. L'articolo 68 non è la licenza di abusare, non è l'impunità. Siamo qui a decidere se poi ci devono essere azioni giudiziarie o no.

l'immunità e l'impunità, ma c'è la possibilità di esprimere delle opinioni, della quale anch'io mi avvalgo ogni tanto, e poi si può essere d'accordo o meno. Oggi la senatrice Rossomando ha dato un'interpretazione, definirei esemplare dell'articolo 68 in riferimento alle vicende della nostra capogruppo Bernini, dicendo che non condivide quelle opinioni, ma sono - viva Dio - delle opinioni di un dibattito che si svolge nel Paese sulla giustizia e quant'altro. Pertanto, prima di spogliarci della nostra libertà di pensiero, riflettiamoci bene, cari colleghi.

Sento anche di dover formulare un ringraziamento sia al presidente Gasparri, sia agli altri colleghi della Giunta, perché più volte ci siamo trovati a discutere di questa materia, il cui contenuto è oggettivamente complesso e merita ancora degli approfondimenti. In questo senso ci siamo lasciati anche l'ultima volta che ne abbiamo discusso. Ribadisco che si tratta di una materia molto delicata e abbastanza complessa e il presidente Gasparri ha inquadrato benissimo l'intera vicenda. Ci impegniamo perché tutto rimanga sempre nei binari della legalità. Credo che la proposta formulata risponda a questi requisiti e quindi il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta del relatore, ma non posso esimermi dall'esprimere in quest'Aula tutte le mie perplessità per la vicenda nella quale è stato coinvolto il senatore Giovanardi; una vicenda che per chi lo conosce e per chi fra i colleghi la voglia approfondire è davvero inquietante e molto preoccupante, in relazione all'invadenza veramente senza precedenti che una certa magistratura ha esercitato nei confronti di un parlamentare che stava svolgendo un ruolo istituzionale, avvera di garantire ciò che a suo giudizio era necessario fare per ristabilire un comportamento equo e rispettoso della legge nei confronti di un imprenditore. Per questa attività, il senatore Giovanardi è accusato davanti a un tribunale di gravissimi reati come rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, violenza e minaccia a un corpo politico amministrativo o giudiziario, oltraggio a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e addirittura originariamente era accusato dell'aggravante mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Penso che chiunque di voi abbia voglia di riflettere per un istante sulla vicenda così come è stata ricostruita dal senatore Malan e dal senatore Gasparri e così come risulta chiaramente dalla lettura della relazione, qualche domanda se la debba porre. Accetto le conclusioni della relazione, secondo cui non vi sono elementi per affermare il *fumus persecutionis*, per quanto - ripeto - da ciò che ho detto qualche dubbio mi sorge quindi non vi sono ragioni per opporsi alla concessione dell'utilizzo dei tabulati telefonici richiesti

è un fatto che ci dovrebbe far riflettere. Per quanto riguarda la richiesta di utilizzazione delle telefonate, va bene concedere la prima, perché si può ancora immaginare che potesse essere occasionale, e certamente respingere tutte le altre, perché essendo molto posteriori, dal 30 marzo della prima all'8 giugno della seconda, è chiaro che il tempo trascorso deve lasciar immaginare che l'autorità giudiziaria sapesse benissimo in realtà chi stava intercettando. È una vicenda di cui il Senato dovrà tornare a occuparsi e che ci deve far molto preoccupare per il confine sempre più labile che l'autorità giudiziaria pensa di spostare sempre in avanti nei rapporti con la politica. Signor Presidente, ovviamente la vicenda è complessa. Abbiamo avuto modo di occuparcene e ce ne occuperemo ancora, con tutta l'attenzione che il caso richiede. Visto, però, che si è ritenuto di intervenire, anticipando anche alcune considerazioni sulla complessità della vicenda, mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, un lavoro all'altezza del compito che ci viene assegnato, cioè quando discutiamo di prerogative garantite dalla Costituzione, ovviamente nel reciproco equilibrio tra poteri dello Stato e nel rispetto, che giustamente rivendichiamo, per l'autonomia della politica. Bisogna avere una coerenza, altrimenti si rischia di essere deboli nelle richieste. Cominciamo, allora, a distinguere. Noi oggi stiamo discutendo e voteremo una relazione, approvata a maggioranza, sull'utilizzo di intercettazioni, che non possono che essere fatte su utenze terze, che indirettamente coinvolgono un parlamentare, e sulle quali, infatti, operiamo una selezione molto rigorosa, secondo i principi che ormai avrete imparato nel corso della giornata odierna. Questa è una prima questione. La seconda questione è che è venuta alla nostra attenzione una registrazione che tecnicamente si chiama registrazione tra privati. Qual è il problema? Ormai secondo la giurisprudenza le registrazioni tra privati possono eventualmente essere acquisite, perché vengono considerate documenti. Stiamo parlando di privati, però. Qui si pone un problema interessante, perché, mentre la norma tutela, comunque, delle forme di registrazione fatte da autorità giudiziaria secondo le modalità che abbiamo detto, c'è

con autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Questo è un argomento che sarà interessante affrontare e, se lo svolgeremo bene, forse sarà utile anche come precedente. Ultimo punto, di non poco rilievo. Ricordiamo sempre che, quando affrontiamo il tema della insindacabilità intesa come opinioni, noi rimaniamo sul piano delle opinioni. L'autorizzazione a procedere *tout court* è stata abrogata. Si può discutere se sia il caso di reintrodurla, alla luce delle considerazioni che ho sentito oggi in Aula. Si può discutere assolutamente di tutto, ma se vogliamo fare un qualcosa di utile, non solo per il caso concreto, ma per le altre questioni che seguiranno, noi dobbiamo ricordare che consideriamo delle condotte, ci vengono rappresentate delle condotte materiali. Pertanto, ci occuperemo con molta attenzione, perché il caso è particolare e complesso, di tutto quanto è ascrivibile all'unica condotta che noi possiamo prendere in esame oggi, che è quella riconducibile ai voti espressi in Aula. che ci sia un'ampia e copiosa attività parlamentare sul tema, ovviamente, è da utilizzare, ma con riferimento a questo. Dovremo analizzare

Se qualcuno vuole farsi fautore di riproporre l'autorizzazione a procedere ampia, è un argomento interessante, che da molti è affrontato ed è anche oggetto di una riflessione dei rapporti tra il potere politico e il cosiddetto controllo di legalità, fin dove possa spingersi, anche alla luce di

fuorvianti, perché rivendicare l'autonomia dell'azione politica e delle battaglie che si possono fare è bellissimo, ma anche poco impegnativo. Poiché l'argomento è molto serio, richiamerei a questo tipo di serietà; perlomeno noi lo stiamo esaminando con grande attenzione e con questo tipo di serietà, facendoci anche carico di fare rilievi giusti e doverosi, a noi non sono arrivati i documenti che eventualmente dovevano pervenire, nelle modalità in cui dovevano arrivare. Non abbiamo mancato e non mancheremo

coinvolti. Fatte queste considerazioni, tornando all'argomento di cui ci dobbiamo occupare, la relazione è molto equilibrata, puntuale e attenta, pertanto il voto del Gruppo PD sarà favorevole.

se esprimerci a favore della deliberazione della Giunta sull'utilizzazione di una intercettazione che evidentemente è stata occasionale e su questo ci dobbiamo confrontare Abbiamo ampliato il dibattito oltre ogni misura, perché naturalmente il senatore Giovanardi ha fatto parecchie audizioni, continua

da parte del senatore Giovanardi, occorre precisare che nel caso di specie il senatore è indagato per il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, violenza, minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e ai suoi singoli componenti, ipotesi aggravate, nonché per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La rivelazione di segreto d'ufficio non è in alcun modo riconducibile al reato di opinione,

questo reato non è ontologicamente un'opinione, ma è qualificato in maniera diversa. Il problema può porsi, semmai, per l'oltraggio,

quindi non trasmetta il tema alla Camera competente per la relativa decisione, allora si può promuovere un conflitto di attribuzione. Tutto questo, però, non è avvenuto, quindi non fa parte dell'attuale decisione che l'Assemblea deve prendere. Si è parlato addirittura di *fumus persecutionis* per quanto riguarda le intercettazioni. Ebbene, le intercettazioni o sono casuali, e allora vanno valutate per la loro occasionalità, quindi non ci può essere *fumus persecutionis* in qualcosa di accidentale, oppure sono indirette o dirette e allora ci vuole l'autorizzazione. il problema del *fumus persecutionis* non può essere affrontato in questa sede e rispetto al tema sottoposto alla nostra valutazione. Pertanto, decidendo sul profilo inerente all'attuale delibera

nel senso di accogliere quindi la richiesta per una sola telefonata, quella iniziale, quella occasionale, quella accidentale del 30 marzo 2013, e di respingerla correttamente correttamente e coerentemente con tutte le successive telefonate che avrebbero potuto indirizzare l'indagine verso tutti coloro che avevano contatti su quel tema con

Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole sulla deliberazione della Giunta delle Grazie infondata l'azione che è stata e che viene portata avanti contro Carlo Giovanardi che, utilizzando quella singola

comprende quanto infondata sia e, anzi, quanto sia ingiusto, come ho detto precedentemente, che un parlamentare debba affrontare le spese, la sofferenza, la cattiva fama che un'azione giudiziaria nei suoi confronti comporta. Sappiamo che questo non è un caso isolato. Io ho sentito parlare

Ora questo non c'è più, ci sono delle residue garanzie, ma è chiaro che, se vengono messe in discussione per ragioni di convenienza elettorale veramente di basso livello, allora il problema c'è.

di chi ha il potere esecutivo. Noi invece siamo un Paese democratico, come tanti altri, per cui c'è questa garanzia. Questa garanzia deriva dalla concezione alla base delle democrazie moderne, cioè che non esistano categorie - pensa un po' - infallibili. Se ci fossero categorie infallibili e perfette, le individueremmo ed esse comanderebbero; non c'è problema, se sono infallibili e perfette saremmo a posto. Se i magistrati fossero perfetti e infallibili si darebbe loro tutto il potere; si abolirebbero il Parlamento, le elezioni e tutte queste cose lunghe e fastidiose (per qualcuno)

accade che in tutte le categorie ci possa essere, accanto ai tanti che si comportano bene, qualcuno che si comporta male. decisione la presero i Padri costituenti nel 1946, nonostante la magistratura, durante il fascismo, avesse generalmente resistito alle pressioni del regime per emettere sentenze orientate politicamente, per la loro dignità, al punto che il regime, per ottenere determinati tipi di condanna, aveva istituito i tribunali speciali. Per questo nella nostra Costituzione il procedimento non può essere sottratto al giudice naturale: tutti principi che dovrebbero essere connaturati in chi si assume la responsabilità di fare il parlamentare. Invece qualcuno ha pensato di andare in direzione opposta.

tra i politici e anche tra i non politici. Tra i non politici è una sanguinosa ingiustizia, che dovrebbe essere la priorità da affrontare quando ci si occupa dei problemi di giustizia. Ogni anno,

Poi ci sono gli altri problemi della detenzione in condizioni non conformi alle norme del diritto internazionale. Questa dovrebbe essere la priorità; altro che approvare il processo eterno, le intercettazioni dappertutto, anche in camera da letto e in ogni circostanza. Questa doveva essere la priorità. Restando all'aspetto politico, se un politico viene distrutto nella sua carriera è un danno alla democrazia e non un danno a quel singolo politico. non si può parlare di rinuncia alle prerogative dell'articolo 68: non è una difesa della persona, ma una difesa della democrazia. *(Applausi)*. Un parlamentare deve poter esercitare il suo mandato senza condizionamenti esterni.

non di Forza Italia stranamente, ma del Partito Democratico, che è stato colpito da decine e decine di cause giudiziarie. E se il parlamentare non può avere questo minimo di garanzia, garantita da quel che resta dell'articolo 68 della Costituzione, vuol dire che deve usare tutto il tuo tempo e tutti i suoi soldi - anzi, più dei soldi che ha - per difendersi nei processi, anziché fare il suo dovere, vale a dire difendere l'interesse dei cittadini italiani. *(Applausi)*. Se non si ha coscienza di questo, forse bisognerebbe fare un altro mestiere, non venire a fare il parlamentare, che è una missione. Difendiamo le dei cittadini qui, perché se il cittadino sceglie una certa persona per rappresentarlo in Parlamento e poi questa certa persona non può fare una cosa perché ha paura che il magistrato lo indaghi, non può farne un'altra perché ha paura che gli facciano causa per diffamazione e deve sopportare decine di conseguenze quindi, non può più vivere né materialmente

Signor Presidente, vorrei che i colleghi che ancora non hanno approfondito con cura la questione della quale ci stiamo occupando sospendessero per qualche secondo l'uso del telefono e si concentrassero su quanto stiamo per votare. Siamo davanti a una vicenda che potrebbe accadere a ciascuno di noi in quest'Aula. Siamo davanti a un senatore, il senatore Giovanardi, che ha ricevuto una segnalazione dal suo territorio. per i parlamentari che non fanno attività di territorio, perché sembra quasi sia vietato e sia necessario stare a Roma tutta la settimana, questo può sembrare anche balzano. Ma noi rappresentiamo territori ed ascoltiamo quanto la gente dice sui territori. Il senatore Giovanardi ha ricevuto una segnalazione dal suo territorio da parte di un'azienda era stata esclusa dalla *white list* per motivi incomprensibili. Che cosa fa un parlamentare eletto dal popolo e rappresentante di un territorio? Si attiva Si attiva in tutte le sedi e con le modalità a lui possibili. E quindi che cosa ha fatto il senatore Giovanardi? Ha fatto quello che tutti coloro che qui cercano di esercitare il mandato con una certa dignità farebbero domani mattina, e cioè si è mosso nella Commissione parlamentare antimafia per modificare le interdittive antimafia; ha presentato atti di interrogazione; si è mosso sul territorio chiedendo alle autorità competenti, quindi al prefetto, al comandante dei Carabinieri e ai vari responsabili degli uffici

il procedimento penale di cui ci stiamo occupando oggi. Vorrei ricordare a chi in quest'Aula, anche stamattina, ha detto che alla fine è inutile che applichiamo l'articolo 68, perché tanto ci sono i giudici che decidono e che basta presentarsi davanti ai giudici con la massima fiducia e poi saranno i magistrati a decidere, che il che il processo è già di per sé molto spesso una punizione, soprattutto per chi è innocente. E se i Padri costituenti hanno immaginato di garantire al parlamentare di poter esercitare tutto il suo mandato, senza limiti o impedimenti che ne vadano a limitare la capacità di azione, è proprio perché questo deve essere posto come bilanciamento tra poteri dello Stato. I poteri dello Stato debbono essere bilanciati, altrimenti - come ha detto poc'anzi il senatore Malan - tanto varrebbe fare il governo dei giudici: fanno tutto loro e noi andiamo a casa. A chi sostiene che bisogna presentarsi serenamente davanti ai giudici e che poi loro sono bravissimi a decidere, chiedo perché

a comprendere come il nostro sistema abbia bisogno delle garanzie di cui all'articolo 68, altrimenti questo Paese finisce nel disastro. Questo è quanto vi dico: fatevi processare, rinunciate alle garanzie, anziché nascondervi dietro al voto, che tanto più o meno, bene o male, la Lega, più Fratelli d'Italia, più Forza Italia, più Partito Democratico ci salvano. Questo vi dico. Tornando nel merito, c'è un equilibrio tra poteri dello Stato che non può essere messo in crisi da qualcuno che usa la cultura del sospetto per gettare ombra, per gettare fango, per usare l'argomento giudiziario nella lotta politica. Questo è quanto sta accadendo al senatore Giovanardi ed è questa la ragione per cui noi voteremo a favore di questa relazione, anche se non è finita. Non è l'ultima parola. Su questa vicenda questa stessa Assemblea dovrà tornare nuovamente, perché non ci sono solo le intercettazioni di cui parliamo oggi, ma ci sono altre questioni che ci riguarderanno. Mi chiedo

forse poteva anche apparire che ci fossero delle pressioni indebite, ma stiamo parlando di condotte tenute dal senatore Giovanardi alla luce del sole, di condotte tenute in questa stessa Aula. Allora significa che noi diventiamo processabili e condannabili per condotte tenute in quest'Aula. Allora diciamo Allora diciamo che noi siamo in libertà provvisoria, finché non troviamo qualcuno che a un certo punto decide di chiuderci la bocca con un processo, com'è accaduto anche a Matteo Salvini in questi giorni,

Potevamo capirlo da soli, non c'era bisogno del tribunale di Catania. Questo è quello che sta accadendo. Guardate che arriva il reddito di cittadinanza, tranquilli; ce n'è per tutti. Fate la domanda che arriva. Torno alla conclusione del mio ragionamento. Siamo di fronte a intercettazioni che, per la loro stessa natura, non sono ammissibili, e giustamente il relatore Durnwalder le dichiara inammissibili. Mi dovete spiegare,

viene sempre intercettato qualcuno con cui il parlamentare stava parlando e, guarda caso, non si fa una sola intercettazione ma ne chiedono 25 da autorizzare. Dico io: una può essere essere casuale, ma se addirittura, come in questo caso, nella prima intercettazione il senatore Giovanardi dice «ci risentiamo a breve»,

Forse viene il dubbio - qualcuno che sedeva in quest'Aula molto più importante, più saggio e anche molto più ironico di me, diceva che a pensar male si fa peccato, ma qualche volta s'azzecca - che in fondo tutti noi siamo costantemente sotto controllo, e a un certo punto, casualmente, arriva la richiesta di autorizzazione di intercettazioni. Ma allora siamo costantemente sotto controllo? Allora c'è qualcuno che ascolta le nostre telefonate e le tira fuori al momento opportuno? Da parlamentare lo voglio sapere; da parlamentare, e prima ancora da cittadino, lo voglio sapere. Voglio sapere se le mie conversazioni sono libere, come prevede la Costituzione, prima ancora che l'articolo 68

e al momento opportuno sarà tirata fuori. A me interessa saperlo; a voi non interessa? Per carità, niente da nascondere, le mie telefonate potrebbero essere tutte pubblicate, ma siamo sicuri che questo sia un buon modo di portare avanti la democrazia?

di espressione e di corrispondenza dei parlamentari sono temi che a mio avviso andrebbero discussi nuovamente.

Colleghi, è intervenuto il senatore Pillon, ora interviene la senatrice Evangelista. Ho richiamato il mio Gruppo, ora richiamo voi; quindi, massima imparzialità. Prego, senatrice. Presidente, effettivamente sul caso Giovanardi mi sembra che si sia sforato ampiamente; addirittura siamo arrivati fino al caso Gregoretti che - vorrei ricordare al senatore Pillon - è stata la Lega a portare in Giunta per martirizzare Salvini in occasione delle elezioni regionali. *(Applausi)*. Sono stati loro a mandare Salvini alla magistratura, quindi il suo stesso partito. Ma torniamo al caso Giovanardi che ci interessa.

il senatore Giovanardi è accusato di aver fatto pressioni a organi politici e a pubblici ufficiali, quindi gli sono contestati diversi reati: rivelazione del segreto d'ufficio, oltraggio, minaccia: il tutto per avere tutelato un'impresa (l'impresa Bianchini) esclusa dalla *white list,* ma che è finita anche sotto processo tanto che alcuni componenti di questa famiglia sono già stati condannati. Ma questo è il merito e il merito non ci doveva interessare, perché la Giunta si doveva occupare solo della richiesta dell'autorità giudiziaria di autorizzazione o meno all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche di conversazioni di terzi a a cui ha partecipato Giovanardi, nonché dell'autorizzazione all'utilizzo di tabulati telefonici, sempre di terze persone indagate per diversi reati, da cui potrebbero uscire delle conversazioni sempre con il senatore Giovanardi. Ebbene, il MoVimento 5 Stelle su questo ha espresso un parere favorevole in Giunta sulla relazione

la prima intercettazione telefonica può essere autorizzata, anche se la magistratura non aveva chiesto preventivamente l'autorizzazione alla Camera competente, poiché per questa conversazione telefonica e per questa intercettazione c'è l'elemento della casualità e del caso fortuito. Per quell'intercettazione l'autorità giudiziaria probabilmente non sapeva che stava intercettando un parlamentare. Riguardo i tabulati telefonici, anche questa richiesta è stata ritenuta legittima perché è stato escluso il *fumus persecutionis*. Certamente non ci sono ragioni di inimicizia con i magistrati che seguono il processo di Giovanardi e soprattutto, anche in questo, si tratta di atti illegittimi e motivati accuratamente nel dettaglio dall'autorità giudiziaria, che indaga su questo caso da diversi anni. Per tutti questi motivi confermo il voto favorevole sulla relazione portata in Aula da parte del MoVimento 5 Stelle.

con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria. *(Segue la votazione)*.

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla sicurezza nel Mediterraneo alla luce degli ultimi sviluppi». Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio. Signor Presidente, vorrei ringraziare il Senato per l'opportunità di condividere alcune riflessioni sui più recenti sviluppi che mettono a rischio la sicurezza del Mediterraneo, area prioritaria della nostra politica estera. Mi soffermerò principalmente su due temi a seguito delle richieste sollevate anche in quest'Aula: in primo luogo, il riaccendersi del conflitto israelo-palestinese, per poi passare alle prospettive del processo di stabilizzazione della Libia, affrontando anche la questione della zona di pesca e la vicenda che pochi giorni fa ha coinvolto alcuni pescherecci italiani. Prima di affrontare gli eventi drammatici degli ultimi giorni in Terrasanta, vorrei fare una premessa. Quanto sta avvenendo riporta prepotentemente alla nostra attenzione l'estrema instabilità di un'area del mondo vitale per la nostra sicurezza, una regione che resta solcata da conflitti regionali e da pericolosi focolai di tensione. Oltre agli avvenimenti in corso in Israele e nei territori palestinesi, pensiamo alla Siria, allo Yemen, all'Iraq, al faticoso percorso di normalizzazione in Libia o alla drammatica situazione economico-sociale del Libano. Come Paese che si proietta nel Mediterraneo quale ponte naturale tra l'Europa e il vicinato meridionale, l'Italia sente particolarmente l'esigenza di elevare l'impegno della comunità internazionale in questo quadrante, con due obiettivi: contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti aperti e, soprattutto, costruire un'agenda positiva per il Mediterraneo che ne valorizzi il potenziale quale piattaforma di connettività tra Europa, Africa e Asia, e quale luogo di collaborazione e prosperità. Le dinamiche geopolitiche che si riverberano sugli equilibri regionali attraversano oggi una fase di grande incertezza, con uno dei pochi punti fermi rappresentato dal ruolo degli Stati Uniti in questa regione, a partire dagli Accordi di Abramo e passando adesso alla stagione della nuova Amministrazione che sta intensificando la cooperazione e le sinergie con i propri alleati, anzitutto con l'Europa, anche in un'ottica di condivisione delle responsabilità. L'impegno della Farnesina in tal senso è costante e coerente. Proprio ieri ho partecipato, dopo aver incoraggiato l'alto rappresentante, Josep Borrell, a convocarla, alla riunione straordinaria del Consiglio affari esteri dell'Unione europea. Sempre ieri ho avuto, inoltre, una conversazione telefonica con il mio omologo israeliano Ashkenazi e il giorno prima ho sentito il mio collega palestinese Malki. Oltre ad altri incontri con attori di primo piano dell'area, due giorni fa ho anche incontrato, in una visita già programmata da tempo, il ministro iraniano Zarif, al quale, come agli altri, ho espresso forte preoccupazione per gli attacchi in Israele e in Palestina, condannando come inaccettabili i lanci di razzi da Gaza e auspicando, al contempo, una pronta de-escalation. Da questi colloqui ho ricavato la conferma di uno dei punti saldi che guidano la nostra politica estera. Soprattutto in questa congiuntura, una distensione a livello regionale non può che passare per la rivitalizzazione dei processi politici di soluzione dei conflitti e di partecipazione democratica. Lo scenario che affrontiamo oggi in Medio Oriente è purtroppo drammatico. La spirale di violenza registratasi negli ultimi giorni in Israele e nei territori palestinesi testimonia la volatilità di un'area frammentata e polarizzata; una volatilità che è il risultato di nodi irrisolti cui si sommano nuovi vettori di instabilità, non ultimo l'inasprimento delle disparità sociali ed economiche indotto dall'impatto della pandemia. Le ultime settimane sono state segnate da un nuovo crescendo di tensioni in Israele e nei territori palestinesi. Abbiamo visto tutti le immagini degli scontri divampati sulla Spianata delle Moschee e Monte del Tempio e nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. I disordini sono presto degenerati in una *escalation* con il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele, con la dura risposta militare di quest'ultimo. Le vittime sono numerose, anche tra la popolazione civile. Tumulti e tafferugli sono divenuti endemici tra ebrei e arabi in varie città a convivenza mista. La comunità internazionale si è immediatamente mobilitata. L'8 maggio, all'intensificarsi degli scontri a Gerusalemme, il Quartetto per il Medio Oriente, composto da Nazioni Unite, Unione europea, Stati Uniti e Federazione Russa, ha rilasciato una dichiarazione in cui si chiamano le parti alla cessazione immediata delle violenze e all'esercizio della massima moderazione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e il suo coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, hanno lanciato l'appello per un'immediata distensione. L'Unione europea, con varie dichiarazioni dell'alto rappresentante, Borrell, si è espressa più volte e appelli alla calma sono giunti anche dalla Casa Bianca, da Paesi dell'Unione, tra cui tra cui Italia, Francia e Germania, e poi dal Regno Unito, dalla Russia e dai principali attori regionali, tra cui Egitto e Giordania, custode dei luoghi santi di Gerusalemme. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito d'urgenza a porte chiuse il 10 e il 12 maggio e da ultimo il 16 maggio, in una sessione pubblica alla quale sono intervenuti il segretario generale, Guterres, e il coordinatore speciale, Guterres ha assicurato che le Nazioni Unite stanno dialogando con tutti gli attori rilevanti per addivenire a un cessate il fuoco immediato e ha indicato quale unica via per un'uscita dalla crisi la realizzazione di una soluzione a due Stati, negoziata tra le parti e in linea con i parametri internazionali. Il Coordinatore speciale, unendosi all'appello del Segretario generale per una cessazione immediata delle ostilità, ha deplorato l'alto costo in vite umane, soprattutto civili, richiamando tutti al rispetto del diritto internazionale umanitario. internazionale umanitario. L'Italia ha fatto sentire la propria voce esprimendo da subito profonda preoccupazione e i nostri appelli si possono sintetizzare in sei punti: fermare immediatamente il conflitto per prevenire la perdita di ulteriori vite umane. Questa resta la nostra priorità. Esprimo anche in questa sede profondo cordoglio per tutte le vittime e vicinanza e solidarietà alle loro famiglie. E non posso che ribadire l'imperativo di cessare immediatamente il confronto militare in atto, per restituire agli israeliani e ai palestinesi il diritto di vivere in pace e in sicurezza. ferma condanna del lancio di razzi da parte di Hamas, che - lo vorrei ricordare - come Unione europea consideriamo un'organizzazione terroristica affinché gli attacchi missilistici dalla Striscia di Gaza cessino con effetto immediato. Lo ripeto: il lancio indiscriminato di razzi è inaccettabile e ingiustificabile. Riconoscimento del diritto alla sicurezza di Israele: riconosciamo il diritto di Israele di proteggere la propria popolazione civile; evidenziamo allo stesso tempo - come ricordato anche dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dall'alto rappresentante dell'Unione europea, Borrell che l'entità della risposta deve essere proporzionata all'attacco subito, nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale. Quarto punto: avviare misure di de-escalation. Deve essere compiuto ogni sforzo per evitare un'estensione del conflitto. È quindi cruciale che le parti si astengano da ogni atto di violenza, provocazione e incitamento all'odio. Mi riferisco innanzi tutto a Gerusalemme, che deve tornare ad essere città di pacifica convivenza, non di intolleranza né di nuovi spargimenti di sangue. È necessario a tal fine che lo *status quo* dei luoghi santi venga rigorosamente rispettato. Le ostilità di questi giorni hanno poi confermato l'insostenibilità della situazione umanitaria e socio-economica a Gaza: una situazione che va affrontata con urgenza. Quinto punto: sostenere il Quartetto per il Medio Oriente. Tentativi di mediazione sono stati tempestivamente messi in campo da parte del Quartetto. Incoraggiamo tutte le parti a impegnarsi costruttivamente assicurando collaborazione a tali sforzi di distensione. Sesto punto: rilanciare il processo di pace. Gli eventi drammatici di cui siamo testimoni segnano, purtroppo, il riemergere di questioni irrisolte, tra le quali le annessioni, gli sfratti e le demolizioni da parte israeliana, che, insieme all'Unione europea e alle Nazioni Unite, abbiamo sempre condannato. Occorre partire dalle cause profonde del conflitto, che generano un senso di frustrazione che si manifesta sotto forme violente ogni volta che il processo di pace mediorientale conosce uno stallo. Bisogna riportare la questione israelo-palestinese nell'alveo di un processo politico, nella cornice di negoziati di pace tra le parti interessate e attraverso forme democratiche di partecipazione e di espressione del dissenso. Come ho già detto, ho trasmesso personalmente questi messaggi al ministro israeliano Gabi Ashkenazy e al ministro palestinese Riyad al-Maliki nei colloqui telefonici che ho avuto con loro negli ultimi due giorni. Il tema è stato anche al centro del Consiglio affari esteri straordinario di ieri, convocato per discutere della crisi. Siamo convinti che l'Unione europea debba prendere una posizione chiara e unitaria e lavorare per riportare la calma e favorire la prospettiva di un ritorno al tavolo negoziale. Ho sostenuto a questo fine l'opportunità che l'Unione sviluppi un'iniziativa diplomatica proattiva, auspicando che il rappresentante speciale dell'Unione europea appena disegnato per il processo di pace in Medio Oriente, Sven Koopmans, possa recarsi quanto prima nella Regione per contatti diretti con le parti. Sul processo di pace mediorientale la posizione dell'Italia è sempre stata molto chiara e ferma: siamo convinti che sia uno snodo centrale per portare stabilità in tutta la Regione, e siamo altrettanto convinti che la sola via per una stabilizzazione duratura è una soluzione a due Stati, giusta e sostenibile, negoziata direttamente tra le parti, in linea con i parametri stabiliti dal diritto internazionale e dalle rilevanti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Solo così israeliani e palestinesi potranno sperare di vivere un giorno in pace e in sicurezza, gli uni al fianco degli altri, con Gerusalemme capitale di entrambi i popoli. Dobbiamo quindi sforzarci di riportare il processo di pace al centro dell'agenda internazionale per realizzare due diritti: quello di Israele di esistere e vivere in pace e sicurezza; quello del popolo palestinese di avere una propria patria. Come accennavo nella mia introduzione, dobbiamo tener conto di linee di tendenza che stanno cambiando, incidendo sullo scenario regionale. La normalizzazione delle relazioni tra Israele e alcuni Paesi arabi - Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan e Marocco - è una di queste. Abbiamo accolto gli Accordi di Abramo con grande favore, nella convinzione che, avvicinando Israele al mondo arabo, queste intese potranno contribuire alla pace e alla stabilità in Medio Oriente. Ma questo percorso di normalizzazione non può in alcun modo sostituirsi al processo di pace. Siamo certi che il sostegno degli Stati Uniti a una soluzione a due Stati potrà concorrere all'avanzamento di questa visione auspicabilmente sinergica tra i due processi. Quest'ultima ondata di forte violenza rende purtroppo ancora più difficile la prospettiva di ripresa di un dialogo anche minimo tra le parti, una condizione di stallo che - devo dire - ho riscontrato già critica durante la mia ultima visita in Israele e Palestina nell'ottobre 2020. Una volta messe a tacere le armi, sappiamo che la china da risalire sarà molto ripida, ma proprio per questo occorrerà fare ogni possibile sforzo per rilanciare l'attività diplomatica, unica possibile via d'uscita da una situazione fortemente deteriorata. La prospettiva di un processo politico non va, quindi, accantonata, anzi rilanciata. In questo senso, siamo determinati a proseguire il cammino intrapreso nell'iniziativa assieme alla Spagna, per contribuire a riportare il processo di pace al centro degli sforzi della comunità internazionale; rinvigorire l'azione del quartetto e innalzare il profilo, per troppo tempo messo in ombra, dell'Unione europea sul *dossier*. L'idea di un'iniziativa congiunta con Madrid nel processo di pace è nata in occasione del vertice italo-spagnolo del 25 novembre scorso, quando ho concordato con la ministra Gonzales di avviare un'azione comune su due direttrici. La prima è volta a far progredire la riflessione sulle modalità di un intensificato impegno dell'Unione europea, favorendo il raggiungimento di una posizione comune che consenta all'Europa di giocare appieno il proprio ruolo. compito non facile alla luce delle diverse sensibilità tra gli Stati membri, ma continueremo, in tal senso, a lavorare con i nostri *partner* a Bruxelles. La seconda direttrice è quella di sviluppare una serie di consultazioni trilaterali con i principali attori internazionali interessati al processo di pace. Fino ad oggi abbiamo tenuto consultazioni a livello di alti funzionari con Giordania, Unione europea, Stati Uniti, Federazione russa e Marocco e intendiamo proseguire, anche innalzando l'esercizio a livello politico. Il nostro scopo non è creare nuovi formati negoziali. Il Quartetto per il Medio Oriente - lo voglio ribadire - è l'unica piattaforma internazionalmente riconosciuta per la mediazione del conflitto israelo-palestinese. Il nostro obiettivo è, piuttosto, mantenere un dialogo approfondito e regolare con tutti gli interlocutori interessati. Abbiamo deciso di adottare un approccio realistico e pragmatico, concentrando la nostra azione, quando le condizioni lo permetteranno, su due fronti: da un lato, vogliamo preservare sul terreno la fattibilità di una soluzione a due Stati, scongiurando ulteriori annessioni di fatto, demolizioni e sfratti da parte di Israele, che sono azioni contrarie al diritto internazionale. In quest'ottica, rimane forte la nostra preoccupazione per il rischio di sfratto al quale restano esposte le famiglie arabe residenti nel quartiere di Sheikh Jarrah e in altre aree di Gerusalemme Est. Vorrei sottolineare che anche la stessa Corte suprema israeliana ha bloccato l'esecuzione degli sfratti per trenta giorni, fino al prossimo 9 giugno. Con l'Unione europea e i *partner* internazionali continueremo a portare avanti un'azione che crei progressivamente le condizioni per misure volte a creare un clima di fiducia tra le parti, misure che continueremo a sostenere anche insieme alla Spagna. Dall'altro lato, intendiamo rilanciare il processo elettorale e la riconciliazione palestinese: elementi essenziali per il consolidamento delle istituzioni e per il rafforzamento della loro legittimità e credibilità internazionale, anche in vista di un ritorno al tavolo negoziale con Israele. È noto come le profonde divisioni interne tra palestinesi abbiano fortemente indebolito la loro credibilità ai tavoli internazionali. Il rinvio delle elezioni da parte dell'Autorità nazionale palestinese, che avrebbero dovuto svolgersi dal 22 maggio, dopo oltre quindici dalle precedenti elezioni nel 2006, ha spinto la popolazione palestinese a mobilitarsi e ha fatto perdere enorme credibilità alle istituzioni della Palestina. Il nostro auspicio è che, non appena le circostanze lo consentano, si definisca un nuovo calendario elettorale e continueremo a sostenere questo processo affinché si creino tutte le condizioni per lo svolgimento delle consultazioni elettorali anche a Gerusalemme Est. Sempre nel Mediterraneo, la Libia è uno dei fronti di instabilità su cui resta la massima attenzione dell'Italia. Il nostro impegno a sostegno della stabilizzazione del Paese è stato e rimarrà costante. Tra le priorità di politica estera e sicurezza nazionale è quella più urgente e delicata. Grazie all'azione della comunità internazionale e delle Nazioni Unite, cui l'Italia ha sempre contribuito attivamente, oggi la Libia, guidata da un'autorità transitoria unificata, è finalmente impegnata in un percorso di transizione istituzionale che troverà compimento nelle elezioni, auspicabilmente entro fine anno. Dopo anni di conflitto interno che hanno stremato la popolazione civile, abbiamo accolto con favore l'avvio di un processo fondato sul dialogo, sempre sostenuto dall'Italia, il raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco e finalmente la designazione di un Governo unificato. Sono passaggi cruciali nel percorso verso la piena stabilizzazione del Paese. Per la prima volta, dal lontano 2014, abbiamo in Libia un interlocutore politico unico, rappresentativo di tutto il Paese: un traguardo impensabile fino a solo un anno fa, mentre era in corso l'offensiva militare contro la capitale. Questi importanti progressi, però, non devono farci abbassare la guardia. La strada verso la pace e la stabilità resta lunga e complessa. Dobbiamo fare un esercizio di realismo e guardare ai molti passi ancora necessari per una completa e duratura stabilizzazione del Paese. La tenuta delle elezioni nella data prevista dalla *road map* adottata a Tunisi dal foro di dialogo politico libico, l'avvio di un effettivo processo di riunificazione delle Istituzioni nazionali, la piena attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco a partire dal ritiro di tutti i combattenti e mercenari stranieri dal Paese, la ricostruzione e il rilancio dell'economia: queste sono le sfide più pressanti che il Governo di unità nazionale è chiamato ad affrontare. Dopo anni di instabilità e incertezza è essenziale che il popolo libico si esprima finalmente in libere elezioni. Le competenti Istituzioni del Paese devono tuttavia ancora definire aspetti costituzionali, legislativi e organizzativi per permettere la tenuta delle elezioni senza posticipi, prima tra tutti la legge elettorale, senza la quale non è possibile assicurare lo svolgimento delle elezioni a dicembre. È poi essenziale definire il quadro costituzionale che dovrebbe emergere dalle elezioni, la cui definizione spetta alla Camera dei rappresentanti e all'Alto Consiglio di Stato. Molti restano ancora i fattori di dubbio interni ed esterni; attori che ostacolano il processo politico poiché preferiscono il mantenimento dello *status quo*. Rimane inoltre prioritario per il Governo garantire l'erogazione dei servizi essenziali alla popolazione come elettricità ed acqua. In questa prospettiva, anche la mancata adozione del bilancio unificato per il 2021 sta complicando la situazione. In questo scenario, l'accordo sul cessate il fuoco concluso a Ginevra il 23 ottobre 2020, che resta un'assoluta priorità, stenta a trovare concreta attuazione sul terreno. Nonostante la riconosciuta determinazione dei membri della Commissione militare congiunta e il completamento delle operazioni di sminamento dell'area, la strada costiera tra Sirte e Misurata, ad esempio, non è stata ancora riaperta a causa delle resistenze di gruppi armati che la controllano e non vogliono lasciare la zona. Questo a testimonianza di quanto ancora precaria sia la situazione di sicurezza, a cui si aggiunge la perdurante presenza di combattenti e mercenari stranieri che potrebbero alimentare anche un rischio terrorismo. Per accompagnare la Libia in questo percorso l'azione dell'Italia si è svolta lungo due direttrici. La prima è quella di un perdurante impegno a livello internazionale a sostegno dell'azione delle delle Nazioni Unite per la stabilizzazione politica del Paese. La seconda direttrice è quella di un'intensa azione di rilancio a tutto tondo nel partenariato bilaterale per rafforzare le Istituzioni nazionali, nell'obiettivo ultimo di una Libia sovrana unita e territorialmente integra. La visita a Tripoli del 6 aprile del presidente Mario Draghi (la prima all'estero quale Presidente del Consiglio italiano), così come le precedenti missioni di preparazione da me svolte il 21 marzo e, poi, con i Ministri francese e tedesco il 25 marzo, nonché la visita a Roma della Ministra degli esteri libica il 22 aprile hanno perseguito esattamente questo duplice obiettivo. Nello stesso solco si inserisce la prossima missione in Italia del primo ministro libico Dbeibeh prevista per il 31 maggio prossimo durante la quale si svolgerà anche un *business forum* che permetterà ai principali attori economici italiani di interloquire con il Primo ministro libico e diversi membri del suo Governo. Sul piano bilaterale molte sono le iniziative. Abbiamo favorito il rafforzamento della presenza politico-istituzionale italiana in tutte le Regioni del Paese attraverso la riattivazione del nostro Consolato a Bengasi. Sono previsti per il prossimo 26 maggio l'insediamento del nostro console Carlo Batori e l'istituzione di un Consolato onorario a Sebha. La Farnesina ha inoltre avviato le procedure per riaprire un ufficio dell'Agenzia per il commercio estero a Tripoli e per la progressiva riattivazione dell'Istituto italiano di cultura nella capitale libica. La nostra azione ha inoltre avviato progetti che erano previsti dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione italo-libico del 2008 e la ripresa dei progetti infrastrutturali aeroportuali per ripristinare e favorire i collegamenti aerei interni in prospettiva con l'Italia. Tra gli altri ambiti in cui si sta sviluppando quest'azione, segnalo la cooperazione sanitaria, culturale, universitaria, in materia di difesa e in campo energetico. A tal proposito, ringrazio tutti coloro della Farnesina che ci hanno lavorato, in particolare l'ambasciatore Pasquale Ferrara, inviato speciale per la Libia. A livello internazionale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sottoscritto e votato all'unanimità due risoluzioni che fotografano la situazione del processo di pace in Libia. Il 23 giugno a Berlino si terrà la conferenza ministeriale per dare ancora più impulso al coordinamento internazionale. Arriviamo ai nostri pescatori. Si evince dalla mia esposizione che, nonostante i progressi politici di notevole importanza, la situazione sul terreno resta ancora fortemente incerta sul piano della sicurezza. Ne è testimonianza anche la difficoltà del primo ministro libico Dbeibeh nel recarsi a Bengasi, due settimane fa, dal momento che gli è stata negata l'autorizzazione all'atterraggio. In questo contesto si inseriscono gli eventi del 6 maggio scorso al largo di Misurata, che hanno coinvolto alcuni pescherecci italiani, tra cui l'"Aliseo". Questo brutto episodio ha rilanciato in maniera drammatica il tema della progressiva territorializzazione del Mar Mediterraneo e delle condizioni di sicurezza. L'incidente è avvenuto a circa 35 miglia dalla costa libica, a nord di Misurata, quando il gruppo di nove imbarcazioni italiane, impegnate nella pesca del gambero rosso, è stato raggiunto da una motovedetta libica in attività di polizia marittima.

e hanno rapidamente assunto una rotta di allontanamento dalla zona. Allo scopo di fermare uno dei pescherecci del gruppo, la motovedetta libica ha aperto il fuoco, con armi portatili, in direzione di "Aliseo", colpendone la plancia e alcune sovrastrutture e provocando ferite, fortunatamente leggere, al comandante. Vorrei sottolinearlo ancora una volta, e lo abbiamo chiaramente detto alle autorità libiche: consideriamo inaccettabile che una loro unità abbia sparato contro le imbarcazioni italiane, esplodendo numerosi colpi che avrebbero potuto avere conseguenze ben più drammatiche per i nostri marittimi. L'arrivo sulla scena della fregata "Libeccio", il cui comando ha potuto interloquire direttamente con quello della motovedetta libica, ha scongiurato ulteriori azioni di forza. Non solo. I contatti contestuali della nostra ambasciata a Tripoli con le autorità locali hanno evitato il sequestro del peschereccio e del suo equipaggio e il rischio del ripetersi della vicenda, drammaticamente nota, che aveva condotto, lo scorso 2 settembre, 18 marittimi di Mazara del Vallo a una detenzione di oltre tre mesi e al sequestro di due pescherecci. Anche l'episodio del 6 maggio, di estrema gravità, testimonia ancora una volta che la zona al largo della Libia in cui operano i nostri pescherecci è molto pericolosa. In almeno altre tre occasioni, negli ultimi due anni e mezzo, vicende analoghe sono state risolte, impedite o prevenute solo grazie a interventi tempestivi del corpo diplomatico a Tripoli o di un'unità della nostra Marina militare in pattugliamento nell'area. Si tratta di una zona che il Comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ha definito, già dal 20 maggio 2019, con una misura tuttora in vigore, ad alto rischio per tutte le navi battenti bandiera italiana, senza distinzione di tipologia (infatti sconsigliamo di andarci). A più riprese tale rischio era stato segnalato dal Ministero degli affari esteri, da ultimo anche con una lettera del capo dell'Unità di crisi al sindaco di Mazara del Vallo, dal Ministero delle politiche agricole, dalla Guardia costiera e dalla Marina militare. La pericolosità non discende solo dalla situazione di conflitto che per diversi anni ha caratterizzato la Libia. Le aree dove si recano i pescherecci in questione si trovano infatti all'interno della zona di pesca protetta proclamata dal Paese nel febbraio 2005. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che sul punto riprende il diritto internazionale consuetudinario, riconosce allo Stato costiero la facoltà di dichiarare unilateralmente una zona economica esclusiva, che può estendersi fino a 200 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale, prevedendo tuttavia che il limite esterno, nel caso di coste opposte adiacenti a quelle di altri Stati, sia definito con accordo, sulla base del diritto internazionale, al fine di raggiungere una soluzione equa. Nella prassi, molti Stati hanno esercitato questa facoltà in modo parziale, mediante l'istituzione di zone di minore ampiezza o di godimento di un numero limitato di diritti sovrani. Queste più specifiche zone non sono espressamente contemplate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ma è pacifico che siano a essa conformi. È dunque di per sé legittima la proclamazione della zona di pesca protetta da parte libica. L'Italia aveva espresso riserve formali sulla proclamazione libica, per il tramite della Presidenza britannica e tedesca dell'Unione europea, nel 2006 e nel 2007; nostre osservazioni si erano concentrate essenzialmente sulla chiusura del Golfo della Sirte e non sulla legittimità della zona di pesca protetta in sé. Dico questo, signor Presidente e signori senatori, perché in questo momento potrei lanciare la sfida dall'altra parte e dire che quelle acque sono nostre, ma da Ministro della Repubblica esporrei i nostri pescherecci, starei segnalando loro di continuare ad andare in quelle acque a rischiare la vita dei nostri uomini e delle nostre donne e questo non lo farò. Avvieremo tutti i processi per negoziare un accordo con la controparte libica, favoriremo le interlocuzioni tra le marinerie libiche e quelle italiane, favoriremo e patrocineremo tutti gli accordi tra soggetti privati, per permettere, bilateralmente, di pescare in quelle acque. Chi oggi dice ai nostri pescatori di andare lì, perché sono acque anche nostre, li sta esponendo, a costo della vita: l'abbiamo visto più di una volta in questi anni. Ci sono due iniziative, che abbiamo avviato nell'ultimo anno e in particolare negli ultimi mesi, con il nuovo Governo. luogo, quando c'è stata la visita della ministra degli esteri al Mangoush qui in Italia, qualche settimana fa, abbiamo avviato un processo per negoziare un accordo sulle delimitazioni marittime. Su questo, signor Presidente,

Se avremo la possibilità di godere di questo nuovo strumento normativo, saremo in grado di compiere le azioni che fanno altri Paesi. Devo però essere molto onesto: l'accordo con la Grecia, simile a quello di cui stiamo parlando, in cui si è riconosciuto il diritto storico dei nostri pescatori, l'Italia ha impiegato venti anni per negoziarlo e l'abbiamo chiuso un anno fa. Quindi non possiamo dare false speranze ai nostri pescatori, però li dobbiamo aiutare ed è per questo che, con il ministro Patuanelli, stiamo per convocare un tavolo,

Non si tratta, come ha detto qualcuno, di dar loro dei sussidi, ma di aiutare un settore economico, che in questo momento ha tutto il diritto di rivendicare la difficoltà in cui si perché oltre alla pandemia si aggiungono le difficoltà di una pesca, che in alcune acque ormai non vede più fauna marina e dall'altra parte, invece, vede la possibilità di andare a pescare. Si tratta di persone, padri e madri di famiglia, che ogni giorno si alzano per andare a lavorare e che hanno tutto il mio e il nostro rispetto. Dobbiamo aiutarli nelle sedi giuste, ma non mettendo a repentaglio la loro vita e quindi la Farnesina continuerà a sconsigliare l'accesso in quelle acque, finché non avremo raggiunto un accordo all'altezza della situazione. Voglio dire un'ultima cosa e poi mi zittisco: non voglio scaricare su qualcun altro le responsabilità. Il tema è tanto drammatico, quanto semplice: negli ultimi dieci anni non c'era neanche un Governo unitario con cui provare a fare un negoziato, per decidere di chi fossero quelle acque. Adesso abbiamo un Governo unificato, ma un processo di pace ancora in corso, nel quale abbiamo bisogno di portare avanti tutti i passaggi che servono, affinché tutte le parti libiche, sia ad Est che ad Ovest, riconoscano l'eventuale accordo che andremo a firmare. Altrimenti saremo punto e a capo ed esporremo ancora una volta le nostre marinerie. La ringrazio nuovamente, signor Presidente, e resto a vostra disposizione.

signor Ministro, i temi che lei ha affrontato sono molteplici, io voglio iniziare dalla fine ed ed esprimerle la solidarietà e la condivisione per la ricerca di un accordo faticoso che lei sta facendo in ordine alla questione che riguarda i pescatori italiani e gli accordi sulle acque territoriali e le acque in cui sarà possibile esercitare questo diritto di pesca. Noi siamo con lei, non credo che nel Parlamento ci possa essere chi preferisce strumentalizzare il disagio e le difficoltà economiche piuttosto che affrontare costruttivamente questo capitolo.

a capire oggi esattamente la situazione in cui il Governo italiano e noi ci troviamo ad operare. Noi abbiamo delle grandissime responsabilità e quando parlo di responsabilità non mi riferisco in particolare all'Italia, ma come parti di una comunità internazionale abbiamo grandissime responsabilità. Ci siamo illusi infatti in questi anni che il silenzio che aveva avvolto la questione palestinese, il conflitto arabo-israeliano, potesse essere una cosa che risolveva e rimuoveva miracolosamente le questioni sul tappeto. Credo, come tutti voi, un difensore rigoroso del diritto del popolo israeliano a vivere in pace, ma allo stesso modo, colleghi, io non posso dimenticare che la politica ripetuta degli insediamenti, che ha spezzettato completamente la territorialità palestinese, rende esasperante una questione su cui la comunità internazionale ha fatto scendere un macigno di silenzio. Quando nella comunità internazionale non si parla, vuol dire che in qualche modo si è complici della situazione che si determina. A questo aggiungiamo, Ministro, una questione; andiamo veloci, seguendo però l'affresco che lei ha fatto. Lei ha ricordato le sue ripetute missioni; le ho fatto in privato gli apprezzamenti per queste missioni e glieli ribadisco in pubblico, ma non dimentichiamo il quadro che abbiamo di fronte. Il nostro Presidente del Consiglio è andato a Tripoli, c'è stata una polemica con Erdogan, che il giorno dopo ha semplicemente chiamato tutto il Governo libico ad andare a Istanbul. Sostanzialmente ha dato una risposta che era la peggiore che ci potevamo aspettare, una sorta di messaggio subliminale: voi andate là, io li chiamo qua e li chiamo tutti, dalle Forze armate alle istituzioni libiche. Questo però capita perché l'abbandono americano del Mediterraneo ha portato oggi un protagonismo nuovo di Russia e di Turchia. Oggi, Ministro, le voglio dire che l'unica cosa seria che il Governo italiano può fare, al di là delle retoriche, delle condanne o delle questioni giustissime di cui stiamo parlando, l'unica cosa che noi possiamo fare è richiamare gli americani all'assunzione della loro responsabilità. Guardate che è una nemesi storica: ricordo le manifestazioni di chi diceva agli americani «*go home*», «andate a casa». Bene, adesso io dico andiamoli a richiamare a casa perché senza di loro lo squilibrio del Mediterraneo è così forte che un'Europa divisa e debole sul piano della politica estera e della difesa non riuscirà mai a risolverlo. Non vorrei essere nei panni del nostro Ministro degli affari esteri e della cooperazione dico scherzosamente, un apprezzamento o un'offesa, deve decidere lei - si colloca nel solco della migliore politica estera italiana, per cui lei sta facendo quello che nella continuità della politica estera è giusto fare. Le sue mani, però, sono legate da una situazione internazionale per cui, senza l'accordo e la complicità profonda degli Stati Uniti d'America, non riusciremo a risolvere questi problemi. Pensate a cosa capita, lei lo ha detto prima: in questi anni, nel silenzio, Hamas ha fortificato i sotterranei e oggi ha armamenti di razzi di ultima generazione. Guardate la quantità di razzi sganciati contro i civili israeliani. In Israele gli insediamenti continuano nelle zone palestinesi come se niente fosse e in questa vicenda abbiamo una paradossale legittimazione, cioè in Israele stavano facendo un Governo contro Netanyahu, che non sono riusciti a realizzare a causa del fatto che Netanyahu ha approfittato della questione

il popolo esasperato, con Hamas che da questo trae giovamento, come trae giovamento dalla nuova condizione del Mediterraneo, perché viene supportato dal Qatar, dalla Turchia, da altre parti del mondo sunnita. Ebbene, colleghi, davanti a questa situazione non possiamo che sperare che l'Europa, in una nuova concertazione multilaterale con Biden, convinca gli Stati Uniti d'America a svolgere un loro ruolo in quest'area, perché altrimenti saremo incapaci di determinare qualsiasi mutamento sostanziale in quest'area.

non è un problema che vede una parte o l'altra del Parlamento, credo che dobbiamo essere onesti su questo: dobbiamo renderci conto che due popoli esistono ed entrambi hanno diritto a stare in pace, ma entrambi

per la prima volta lo scontro tra arabi e israeliani non è solo nei territori, ma è nelle città israeliane, cioè si è inserito un veleno supplementare che porta discordia e divisione all'interno dello stesso territorio dello Stato d'Israele. Abbiamo tanti elementi di preoccupazione e ricordo che Fanfani, Andreotti, Colombo, ma anche Craxi e le grandi tradizioni repubblicane e socialiste hanno sempre collocato l'Italia a difesa di Israele, ma con grande attenzione alla questione palestinese e al mondo arabo, perché è il mondo che noi compartiamo nel Mediterraneo. Mi auguro, quindi, che nella concertazione di un multilateralismo rinnovato ci possa essere un'iniziativa congiunta fra Europa e America, perché non vedo un'alternativa efficace. Se andremo avanti da soli, rischiamo di essere assolutamente complementari e incapaci di dare un nostro contributo.

L'intervento del senatore Casini mi mette nella condizione di tagliare per lo meno di un minuto alcune considerazioni che volevo fare, proprio perché lo condivido. Mi preme, però, sottolineare due aspetti della sua relazione, signor Ministro, Ministro, perché sono i due poli attorno ai quali si è sviluppata nel tempo la politica estera italiana (sono stati ricordati anche i suoi rappresentanti nel passato, da Craxi ad Andreotti a De Michelis) fino alla alla proposta che lei ha messo oggi sul tavolo: il diritto alla pace e alla sicurezza da parte di Israele, da una parte, e, contestualmente, il diritto del popolo palestinese ad avere una patria certa e certificata. Quello che sappiamo è che, nonostante gli accordi siglati più volte, in ultimo gli Accordi di Abramo, prima ancora quelli di Oslo e poi di Camp David, il conflitto è ripreso. A differenza del passato, poiché lo scenario politico internazionale è cambiato ed è in via di mutamento, quello che sta succedendo, se non riusciamo a far tacere le armi, rischia di non portare nulla di buono. Sul conflitto israelo-palestinese, a differenza del passato, c'è una sorta di danza tribale di potenze regionali, che esercitano su quella stretta di terra il loro potere in divenire. I nomi sono quelli che conosciamo. Li ha fatti anche lei: la Russia, la Turchia e dall'interno l'Iran. La novità è il Governo che fa capo a Erdogan. È un elemento in più. Su questo, io sono molto più pessimista dell'amico senatore Casini sul fatto che l'Europa svolga principalmente una sua funzione senza aspettare l'azione degli degli Stati Uniti d'America e della nuova presidenza Biden. Dico ciò perché quello che sta accadendo è figlio di una storia che dura ormai da oltre mezzo secolo. Non c'è dubbio che sia stato rinfocolato da intemperanze e decisioni sbagliate, che hanno avuto alla testa il precedente Presidente degli Stati Uniti, Trump, ma non c'è altresì dubbio che la politica estera degli americani, fin dal presidente Obama, rispetto all'area mediorientale abbia assunto caratteristiche diverse da quelle di chi ha preceduto Obama alla presidenza americana fino alla tradizione più recente. Quello che sappiamo oggi è che stanno prevalendo, da entrambe le parti, estremismi, gruppi dirigenti poco lungimiranti da parte palestinese e da parte israeliana, ragioni politiche interne che riescono a far prevalere posizioni estreme. Da un lato, c'è un popolo che vive in grandi città, che ha

un muro che incombe su quella che la leggenda narra essere "la mangiatoia del Cristo Redentore". Questa è la fotografia del reale. Non c'è dubbio che l'eccesso di provocazioni sulla Spianata delle Moschee il giorno della fine del Ramadan e poi il lancio dei missili abbiano generato una provocazione; ma non c'è dubbio che quella provocazione sia stata altrettanto esagerata.

va riconosciuto al popolo palestinese il ripristino dei diritti che sono stati lesi. Terzo: bisogna ripartire da ciò che fa diritto internazionale, le risoluzioni dell'ONU, per riconoscere il doppio diritto alla sicurezza nella vita di due Stati. Se il Governo italiano, insieme ai Paesi rivieraschi e mediterranei, riuscirà a svolgere questa funzione, in rapporto stretto con l'Unione europea, avrà preso la strada giusta per l'avvenire.

Sta succedendo una cosa incredibile in questi giorni, perché un'ondata di menzogne sta sommergendo il popolo palestinese proprio mentre è sotto i bombardamenti di uno dei più efficienti eserciti di occupazione coloniale del mondo. Non sono alla pari gli scontri di cui leggiamo ogni giorno, non sono scontri tra due contendenti pari ed equivalenti, non lo sono mai stati. La cosa sconvolgente è che con difficoltà riusciamo a rintracciare accenni di riflessione storica che ci possano ricondurre alla verità. Eppure solo partendo da un atto di verità si può provare a ripartire. L'ultimo rapporto dello Human rights watch del 27 aprile dichiara lo Stato israeliano colpevole di crimini contro l'umanità, crimini di *apartheid* specifica. Ricordo che Human rights watch è, insieme ad Amnesty international, la voce più autorevole, seria e indipendente nel campo dei diritti umani a livello internazionale; il suo giudizio legale è stato redatto in un rapporto di 213 pagine; la pubblicazione arriva all'indomani di due settimane di scontri e violenze a Gerusalemme. Cosa è successo per cui dall'inizio del *ramadan* a metà aprile Gerusalemme è sull'orlo dell'esplosione? Tutto ha avuto inizio durante il mese sacro per l'Islam*:* i palestinesi di Gerusalemme hanno l'abitudine di ritrovarsi la sera nei pressi della porta di Damasco, uno degli accessi alla moschea della città vecchia, ma a metà aprile le autorità israeliane hanno chiuso l'area ai palestinesi. Si tratta di una misura umiliante, applicata senza dare nessuna spiegazione, che ha provocato le proteste dei palestinesi, represse dalla polizia israeliana. Ciò a dimostrare ancora una volta che i cittadini palestinesi non sono considerati cittadini al pari degli altri. La loro stessa presenza non è tollerata, alla faccia dell'integrazione e delle città miste di cui parlano gli occidentali. In realtà sono luoghi di discriminazione, dove si macera la crisi israeliana, che non tollera di avere 7 milioni di palestinesi sul suolo della Palestina storica. Il Covid, ancora una volta cartina di tornasole, ce lo dimostra con i numeri:

come mai, all'annuncio della Santa Sede di voler riconoscere lo Stato di Palestina, il Governo israeliano ha protestato; si risponde Netanyahu non vuole nessuno Stato palestinese. Lo dimostra - aggiunge - la legge che esclude gli israeliani palestinesi dalla piena cittadinanza che viene riservata solo agli israeliani ebrei. Di tutto questo sulla stampa italiana vi è poco o nulla. Tutti si sono concentrati su Hamas, ma essere a favore della Palestina, signor Ministro, non significa essere a favore di Hamas, perché Hamas non è a favore della Palestina, la usa; tuttavia, essere contro Hamas non può in nessun modo voler dire essere con Netanyahu. Chi paga sono sempre i popoli, definitivamente ostaggio del potere politico che avversa ogni soluzione di pace.

l'ultimo teatro del consolidamento di un'occupazione che rende la soluzione dei due Stati sempre più anacronistica e illusoria. Non c'è alcuna equivalenza in questo conflitto sempre più dimenticato dall'opinione pubblica internazionale. Vi è un'abissale asimmetria alimentata da quello che avrebbe dovuto essere il paciere, gli Stati Uniti, che con Trump ha compiuto i passi più significativi nella divisione, decidendo di non considerare le

Eppure i palestinesi di Gerusalemme Est, annessa a Israele sin dal 1967, non sono considerati cittadini, godendo solo di uno *status* di residenti, che può essere revocato in qualsiasi momento. Signor Presidente, signor Ministro degli esteri, colleghi senatori, comprendo e condivido le ragioni dell'allarme diffuso per quel che sta accadendo in Medio Oriente, ma credo non sia inutile, anche avendo sentito quest'ultimo intervento, ragionare anche su quello che sta succedendo da noi, in Occidente. Dunque, il popolo curdo rispetto alla Turchia; le minoranze uiguri, tibetana e mongola rispetto alla Cina; i cittadini di Hong Kong nuovamente rispetto alla Cina; il popolo armeno del Nagorno Karabakh rispetto all'Azerbaijan e quindi rispetto alla Turchia, di fatto; i cittadini venezuelani rispetto al regime autoritario di Maduro; le popolazioni dell'Abkhazia e dell'Ossezia in Georgia; i tamil nello Sri Lanka; la popolazione karen in Birmania... Presidente, potrei andare avanti mezz'ora. Mi auto contengo, ma le assicuro che l'elenco dei popoli in cerca di Stato, delle minoranze - a torto o a ragione - considerate oppresse è sterminato, letteralmente sterminato. Etnia per etnia, religione per religione, lingua per lingua, potrei continuare questo elenco a lungo. E in questo elenco dovrei mettere senz'altro anche i cristiani perseguitati in Somalia, in Nord Corea, nelle nelle Isole Molucche, in Burkina Faso, in Camerun, in Congo, in Nigeria. Insomma, ogni giorno vengono uccisi dai 13 ai 18 cristiani, solo in quanto cristiani. Di tutto questo tendenzialmente le *élite* occidentali non si occupano. Io non vedo manifestazioni di piazza per difendere questi popoli, queste etnie, queste minoranze religiose; non vedo raccolte di firme, non leggo vibranti editoriali, non mi pare che ci siano una quantità di Capi di Stato o di Governo, di *leader* politici, di organizzazioni internazionali dei diritti umani che si fanno carico di queste enormi e immense sofferenze, che sono sotto i nostri occhi, se volessimo vederle. Mi pare che ci sia soltanto un caso in cui le *élite* occidentali si mobilitano con grande passione e coinvolgimento emotivo: il caso del conflitto arabo-israeliano, tra il popolo palestinese palestinese e lo Stato d'Israele, Stato che, secondo Hamas, non avrebbe diritto di esistere. Allora, se la logica ha ancora un qualche spazio tra i nostri ranghi, le possibili spiegazioni credo che siano soltanto due: o esiste una particolare affinità culturale, politica, strategica, geopolitica, religiosa da parte di queste *élite* rispetto ai palestinesi o esiste una particolare ostilità nei confronti dello Stato di Israele. Ora, io sbaglierò ma in tutta sincerità questa affinità non la vedo, non la riscontro; ne deduco, quindi, che il problema è lo Stato di Israele. Ma cosa ha lo Stato di Israele di diverso dagli altri? Qual è lo specifico dello Stato di Israele? Lo specifico dello Stato d'Israele, colleghi, Presidente,

se avessimo il coraggio intellettuale di ammettere che - non sempre, naturalmente, ma nella maggior parte dei casi o comunque molto spesso - l'antisionismo è l'abito buono dell'antisemitismo.

le sirene, la notte illuminata dai missili dei terroristi islamisti di Hamas, l'angoscia di essere colpiti, la speranza che il sistema di difesa entri in azione: questo è quello che provano i cittadini di Israele sotto attacco nelle loro notti. Il bilancio dell'ultima crisi israelo-palestinese conta ad oggi oltre 3.000 razzi lanciati da Hamas contro città e obiettivi israeliani, inclusa Gerusalemme, che è la culla della nostra civiltà. Abbiamo chiesto una ferma condanna anche da parte del Governo italiano per ribadire una lunga vita a Israele, che difende il diritto di esistere nella pace e nella convivenza fra i popoli. pertanto citare alcune parole molto importanti che la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello ha lanciato la scorsa settimana: «Israele è sotto attacco. In questo momento da Gaza piovono missili sui cittadini israeliani». Per questo ha invitato tutti al Portico d'Ottavia, la scorsa settimana, per una manifestazione di vicinanza e solidarietà agli amici di Israele e della pace, perché «Gli amici di Israele e della pace sono i benvenuti». Ecco, queste parole sono, secondo me, molto importanti. Soprattutto, ricordo in quest'Aula che noi c'eravamo al Portico d'Ottavia. C'era la Lega con Matteo Salvini, ma c'erano anche altre forze politiche: c'era Forza Italia con Tajani, c'era il PD con Letta, c'era la Boschi e c'era anche il MoVimento 5 Stelle. C'eravamo tutti il nostro *leader* Matteo Salvini ha anche ricevuto minacce gravissime proprio per questa sua presenza e per le sue affermazioni, e per questo rinnoviamo la solidarietà al nostro Matteo Salvini. Credo che in politica estera occorra anche dire da che parte stare, e noi sappiamo da che parte stare; l'Italia sa da che parte stare, e lei, che è il nostro Ministro degli esteri, sa bene che deve dimostrarlo quotidianamente. Vorrei dire che noi già avevamo fatto una scelta importante con il contratto di Governo giallo-verde - forse qualcuno lo ricorderà - in cui c'era scritto nero su bianco che l'Italia ha un *partner* privilegiato, un amico storico, ossia gli Stati Uniti. il nostro *partner* sono gli Stati Uniti, allora anche lo Stato d'Israele è un nostro *partner* privilegiato e chi attacca Israele attacca noi e anche la democrazia. Purtroppo, devo però segnalare un fatto sul quale siamo rimasti molto sorpresi e cioè che questa settimana è stato in visita qui a Roma Javad Zarif, ministro degli esteri iraniano, di quella Nazione che molti indicano proprio come il vero elemento destabilizzante dell'area mediorientale. L'ambasciatore di Israele a Roma Dror Eydar ha inviato un messaggio durissimo di condanna, attraverso le colonne di un quotidiano, proprio al Ministro degli esteri iraniano, dicendo: «qualunque elemento moderato in Medio Oriente cerchi di attuare la normalizzazione con Israele, voi iraniani lo minacciate». lo minacciate». Noi riteniamo, soprattutto in questo periodo di conflitto così acceso tra le parti, che iniziative che mostrino un atteggiamento di tolleranza verso determinati soggetti quali l'Iran non siano sicuramente da approvare. Non è sicuramente attraverso azioni che fomentano l'odio tra i popoli che riusciremo a risolvere la questione israelo-palestinese. Non è sicuramente dialogando con chi fomenta quell'odio che porteremo finalmente la stabilità in quei territori. degli esteri, sicuramente nelle prossime settimane tornerà alla ribalta una delle possibili soluzioni, che è quella dei due popoli in due Stati. Vedremo se sarà quella la strada e se servirà per risolvere questo conflitto. Sicuramente dovremo mettere allo stesso tavolo interlocutori credibili e riconosciuti, ma sicuramente non è un interlocutore Hamas, che lancia razzi a migliaia contro un popolo sovrano, sapendo che il 20 per cento di quei razzi precipiterà sempre sui palestinesi. Concludo il mio intervento, ribadendo ancora il concetto che in politica estera bisogna saper scegliere da che parte stare; l'Italia lo ha già fatto le sue parole ce l'hanno dimostrato. Lo abbiamo fatto noi tutti insieme anche la scorsa settimana al Portico d'Ottavia, insieme, al fianco di Israele. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci sono tanti ebrei e musulmani che in questi giorni stanno ripetendo: ci rifiutiamo di essere nemici. Ne è un esempio il personale ospedaliero dell'HaEmek Medical Center nella città israeliana di Afula. La stampa internazionale riporta infatti come i medici e gli infermieri di questa clinica, sia arabi sia israeliani, impegnati nel soccorso delle vittime dei bombardamenti, cantino ogni giorno una canzone popolare, «Od Yavo Shalom Aleinu», che in ebraico significa «La pace arriverà ancora»: un canto di buon auspicio, insieme, come appello a che finiscano gli scontri e si ritorni a una convivenza pacifica che in queste ore sembra ancora purtroppo lontana. Tra Israele e Gaza negli ultimi dieci giorni ci sono stati 63 bambini uccisi dagli attacchi, altri 400 sono stati feriti e gli scontri non accennano ancora fermarsi. Oltre 4.000 razzi sono stati lanciati tra Israele e Gaza, almeno 50 sono le scuole danneggiate. Ho volutamente evitato di distinguere quali e quanti razzi siano caduti a Gaza o in Israele, quante scuole siano state distrutte a Gaza o in Israele, o quanti tra i minori uccisi fossero dell'una o dell'altra cittadinanza. Ho voluto evitare di distinguere, perché non è una questione di appartenenza geografica o religiosa. I civili e i bambini che stanno morendo sono un dramma dell'umanità tutta, perché i morti non hanno colore, né religione. Ecco perché ribadiamo che il lancio indiscriminato di razzi e mortai contro i centri abitati israeliani è inaccettabile e, allo stesso modo, diciamo a Israele che il diritto legittimo di difendere il proprio popolo da attacchi terroristici non deve giustificare atti di forza sproporzionati contro la popolazione civile palestinese. Come Italia Viva sosteniamo i tentativi di mediazione di Europa, Nazioni Unite, Stati Uniti e Federazione Russa. L'obiettivo principale dev'essere quello di un immediato cessate il fuoco e di una progressiva de-escalation*,* che porti velocemente a una stabilizzazione, per poi lavorare a una soluzione duratura del conflitto, cioè la previsione di due Stati, così che entrambi i popoli possano vedere riconosciuto il proprio diritto a esistere e ad avere un luogo in cui vivere e dove esercitare pienamente il proprio culto. Infatti, se è vero che il problema tra Israele e Palestina è uno scontro tra religioni, tra ebrei e musulmani, è anche vero che si tratta di un conflitto per gli spazi di sopravvivenza, per la terra. Non a caso, l'elemento scatenante che ha dato origine al lancio di missili di Hamas verso Israele la settimana scorsa è derivato dall'ennesimo tentativo di sfratto a famiglie palestinesi. È una realtà: da decenni Netanyahu è prigioniero dell'estrema destra integralista, che rivendica insediamenti ed espande le proprie colonie a danno di una progressiva emarginazione dei palestinesi. Ecco che, se si vuole tornare a parlare e a lavorare per la pace, questa situazione va fermata. Non bisogna lasciare che siano estremisti a determinare il corso delle cose. Bisogna riprendere il dialogo, così da creare i presupposti per dare concretezza al principio di "due popoli, due Stati", che ad oggi è l'unica soluzione per garantire la pace. Il tentativo degli Accordi di Abramo, stilati nel settembre del 2020 con l'obiettivo di promuovere rapporti privilegiati tra Israele e alcuni Paesi arabi, rischia di non avere sviluppi. Gli attacchi alla Palestina da parte di Israele hanno provocato reazioni di rabbia in diverse piazze del mondo musulmano, anche nei Paesi aderenti agli Accordi di Abramo, i cui *leader* adesso, per sedare le contestazioni, prendono le distanze da Israele, dopo anni nei quali sembrava che il conflitto israelo-palestinese potesse essere accantonato e le istanze palestinesi potessero finire nel dimenticatoio, l'attualità degli attacchi dimostra invece come quel conflitto continui a essere centrale per la soluzione dei problemi mediorientali. Ecco che serve uno sforzo supplementare per pervenire a una soluzione duratura. Senza un accordo politico, non ci sarà pace e noi siamo i primi ad avere tutto da perdere nell'instabilità del Mediterraneo. Pensiamo anche alla Libia, rispetto alla quale è altrettanto essenziale contribuire al processo di stabilizzazione, prodigandosi per legittimare quanto prima la pesca dei nostri pescatori e soprattutto affinché non si verifichino più ulteriori aggressioni nei confronti dei nostri pescherecci. La questione mediorientale è un importante banco di prova, con il quale ci troviamo a misurarci e ha ragione Papa Francesco, che nell'omelia di domenica scorsa ha detto: «Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l'altro?». E poi ha chiesto che si percorra la via della pace. Solo così la canzone della libertà di medici ed infermieri all'ospedale di Afula potrà concretizzarsi in fretta, dimostrando che arabi ed ebrei possono riuscire per davvero a non essere più nemici. Fratelli d'Italia si è configurata in questo Parlamento, e tanto più a confronto di questo Governo, come un'opposizione patriottica e l'opposizione è sempre patriottica, patriottica, in ogni contesto, soprattutto quando si parla di interesse nazionale, quando è in gioco la sovranità nazionale, quando si definisce la politica estera che non riguarda i partiti; riguarda gli Stati, definisce gli Stati e quindi le Nazioni. Per questo, signor Ministro, non si stupisca che Fratelli d'Italia sia oggi, su questi temi, intenta a cercare soluzioni, non a denunciare problemi, ma a trovare la strada per risolverli. Questo vale anche per quanto riguarda i nostri pescatori e il loro diritto a pescare e a lavorare nelle acque internazionali. Questo è tanto vero che,

il 2 novembre dello scorso anno, per definire quale potesse essere la strada che l'Italia avrebbe potuto perseguire per risolvere il problema, che non è soltanto quello delle acque territoriali con la Libia. In quella mozione di dieci punti c'è tutta una strategia che un Paese, una Nazione, dovrebbe attuare in modo unitario e coeso in politica essere per definire i confini marittimi del Mediterraneo. Non è un caso, infatti, quanto sta accadendo nel Mediterraneo: nasce dalla consapevolezza che il futuro dei popoli passa attraverso l'economia delle acque dei mari; perché il Mediterraneo non è soltanto il mare dei pescatori e delle loro famiglie, che dobbiamo sorreggere e proteggere. È anche il mare delle risorse minerarie, energetiche, dell'energia rinnovabile, dei cavi sottomarini; il futuro dei popoli passa negli oceani e soprattutto nel Mediterraneo. Definire i confini marittimi significa attuare una politica che l'Italia, purtroppo, non ha perseguito e che l'Europa non persegue per risolvere i problemi dei confini, che non sono soltanto quelli con la Libia; sono quelli con l'Algeria, con Cipro, con la Slovenia, persino con la Francia, così come con la Croazia. Tutto questo fa parte di una politica che abbiamo definito in Parlamento con un'apposita mozione e vorremmo che di questo si discutesse insieme in un'occasione per definirla e perseguirla, Governo di oggi e quelli di domani, che in questo non si possono confrontare e scontrare, perché sono i Governi della Nazione che attuano la politica estera e l'interesse nazionale, comunque e sempre. Ciò vale per quanto riguarda la questione delle acque per i nostri pescatori, ma vale - e non a caso - per tutto il Mediterraneo, perché nel frattempo che lei è stato convocato qui, signor Ministro, è scoppiato qualcos'altro e altro sta per scoppiare. Il problema è gigantesco e l'Italia è al centro del problema e dei conflitti, perché in Libia oggi non si confrontano più le potenze europee; si confrontano e si scontrano le potenze sunnite con le armi dell'ideologia e spesso anche del fondamentalismo. l'assenza dell'Europa l'ha causato; le divisioni europee hanno condannato la Libia a quello che è accaduto. Lo stesso accade - lo voglio dire con consapevolezza - con stessi interlocutori, in Palestina e in Israele, perché non può sfuggire ad alcuno quello che prima diceva anche il presidente Casini. Dopo la visita di Draghi a Tripoli e dopo che l'Italia è tornata a essere l'alleato atlantico nel Mediterraneo degli Stati Uniti, la Turchia ha riaperto le rotte dei migranti, stavolta non nei Balcani,

E le motovedette oggi sono addestrate dai turchi. Non è un caso che la Turchia abbia alimentato anche quello che sta accadendo a Gaza, perché chi soffia sul fuoco è soprattutto, purtroppo, il regime di Erdogan con cui dobbiamo convivere, ben sapendo che l'Italia ha tanti interessi anche in Turchia, ma ben sapendo anche come quel regime si muove. Ebbene, nella terra della Palestina e nella terra di Israele c'è tutto; non ci sono solo la sofferenza degli ebrei e dei musulmani, ma anche quella dei cristiani, perché Gerusalemme è la città santa per tutti noi e per loro. Tutti noi, in qualche misura, nella nostra storia politica ci siamo illusi di poter fare qualcosa. Io stesso, quando ero al Governo, sono stato tre volte in Israele. Ho incontrato Shimon Peres, Sharon, Olmert

e non dobbiamo rassegnarci a tornare lì, così come purtroppo tutti ci siamo ritrovati, ancora una volta, al Portico d'Ottavia. Quante volte ciascuno di noi è stato costretto o ha sentito la necessità di andare al ghetto, al Portico d'Ottavia, davanti alla sinagoga per dire con forza che tutti siamo a difesa della sicurezza di Israele, anche perché con Israele e con i popoli europei e occidentali condividiamo gli stessi valori di fondo, che sono quelli della civiltà ebraica, cristiana romana. Con gli altri evidentemente dobbiamo confrontarci come *partner*, ma una cosa è condividere i valori ed essere alleati, altra è trattare con gli altri affinché i popoli possano progredire nella pace. Questa certezza ce la dobbiamo dare da italiani, quindi da europei e, di conseguenza da occidentali, quindi atlantici. Ebbene, al Portico d'Ottavia siamo andati tante, troppe volte. tante, troppe volte. Ora bisogna tornare su quella terra e comprendere che, se lì non si risolve quella questione,

perché il processo in Germania rende più debole quello che potrebbe essere il nostro principale *partner* (la Germania) nel contesto mediterraneo. È evidente a tutti che la crisi europea è dei ruoli e la mancanza della politica estera europea, accanto all'assenza degli Stati Uniti in quel contesto, ha determinato la presenza di potenze regionali che confliggono tra di loro per la supremazia nel mondo islamico e non solo, anche per questioni che possono essere territoriali, economiche e dinastiche. Quando c'erano le grandi potenze, regolavano l'equilibrio del mondo. Oggi non ci sono. Il nuovo conflitto globale, di cui dobbiamo essere consapevoli noi più di altri,

la più grande potenza mondiale. Non era mai accaduto, nemmeno durante il periodo dell'Unione Sovietica, che ci fosse questa reale minaccia. Oggi questa minaccia c'è e per questo ci interessiamo sino in fondo del diritto dei popoli a Hong Kong,

Lo possiamo fare oggi più che mai con i nostri *partner* europei e occidentali per avere quel ruolo che è evidente in ciò che stanno facendo i nostri soldati come forza di interposizione nel Libano. Lì le bombe non ci sono, perché ci sono, con il loro sacrificio e il loro coraggio, i soldati italiani.

Parto dalla Libia per poi concentrarmi sul tema principale del suo intervento. Penso che l'Italia si sia mossa per tempo, questa volta, e abbia colto la finestra di opportunità che si è aperta con l'avvento del nuovo *Premier* e con un tentativo di unificazione a cui le diplomazie internazionali lavoravano da tempo. Quindi, bene che l'Europa si muova insieme (e quando dico Europa, in questo caso, mi riferisco al coordinamento delle politiche estere dei principali Paesi, in particolare Francia, Germania e Italia). Siamo stati i principali attori e ricordo le sue visite, ministro Di Maio, e quella del *premier* Draghi, che apre una fase nuova dal punto di vista commerciale e politico.

Colgo l'occasione per ringraziare anche io le donne e gli uomini della Marina militare italiana, che meritano il nostro ringraziamento e il plauso perché, se non è successo ancora ciò che abbiamo visto in passato, è proprio grazie a loro. *(Applausi)*. Penso però che adesso sia nostro dovere dare una definizione per cui non dobbiamo assistere, come in passato, agli accordi fatti da Federpesca, con il Governo che fingeva di non vedere. È giusto dare una risposta a un settore per noi importante, come quello ittico, e definire con la Libia un accordo molto chiaro. Veniamo al tema principale. A nome del Partito Democratico, vorrei piena solidarietà al popolo palestinese e a quello israeliano - sia agli arabi, sia agli ebrei - per i lutti e le sofferenze che continuano a patire, evidentemente per colpa non loro, ma di chi li governa. Voglio sottolineare che il Governo si è mosso nei principali *forum* multilaterali per chiedere immediatamente lo *stop* al ricorso alle armi e il cessate il fuoco. Da questo punto di vista, bene la condanna di Hamas inserita nella lista delle organizzazioni internazionali e basta al lancio indiscriminato di razzi sulle città

Aggiungo un punto. A un Paese con cui abbiamo relazioni politiche e diplomatiche consolidate, a un Paese amico, noi abbiamo il dovere di ricordare con estrema chiarezza la la consapevolezza della propria forza e della propria superiorità militare. Questa sproporzione di forza non può e non deve andare a danno della popolazione palestinese e spesso di civili indifesi.

Assistiamo a una situazione in cui Netanyahu, da dodici anni al potere e alle prese con i suoi guai giudiziari, sembrava poter essere messo definitivamente alla porta della politica israeliana, con il tentativo di Lapid di formare un nuovo Governo. L'emergenza probabilmente anche provocazioni calcolate e studiate hanno riportato Netanyahu al centro della scena e hanno fatto fallire il tentativo di Lapid, che avrebbe portato anche la lista araba unita all'interno della nuova coalizione. Le responsabilità sono evidenti nella Spianata delle Moschee proprio durante il Ramadan, con il simbolismo che in quelle terre è ancora più forte e soprattutto con la provocazione degli sfratti a Sheikh Jarrah. Quello è uno dei principi più delicati: riaffermare il diritto al ritorno in quelle terre martoriate, in cui faticosamente si tentano episodi e sperimentazioni di integrazione; il diritto al ritorno praticato, spinto e tollerato dal governo Netanyahu pone una ferita difficilmente sondabile e un macigno sul progetto dei "due popoli, due stati", di cui spesso la comunità internazionale si riempie la bocca, ma che rischia di diventare una declamazione vuota. Da parte palestinese non ci devono essere alibi, perché anche al-Fatah non può certo dire che sia solo colpa israeliana, che non permetteva il voto all'interno di Gerusalemme Est. È evidente come al-Fatah fosse in crisi di consensi e come fossero addirittura tre le liste presentate, non solo i sostenitori di Abbas (Abu Mazen), ma anche quelli di Barghuthi e quelli di Dahlan, che mettevano in discussione al-Fatah nei confronti di Hamas. Due estremismi, Hamas e il Governo guidato da Netanyahu, che mettono in crisi un processo di pace che si è aperto. L'altro grande tema su cui voglio andare a concludere, ma anche essere estremamente chiaro e attirare l'attenzione di quest'Assemblea,

la debolezza della Russia, non a caso sfidata dalla Turchia nel Mediterraneo, e la debolezza del sistema delle Nazioni Unite, che si è limitato a un appello pilatesco, parlando del diritto di Israele a difendersi e, dall'altra parte, del diritto all'autodeterminazione dei palestinesi. Gli Stati Uniti sono di fatto usciti da tempo dal sistema onusiano, perché i danni fatti da Trump li misuriamo anche in questa vicenda e in questo passaggio, con la debolezza delle Nazioni Unite, orfane degli Stati Uniti, e con la Cina che non a caso cerca di inserirsi e addirittura di ospitare da loro il nuovo *round* di un incontro fra i principali attori palestinesi e israeliani. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ci aspettiamo da Biden un cambio di passo e che ritornino a essere protagonisti nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Gli Accordi di Abramo, rispetto allo stallo che c'era e a una comunità internazionale seduta sul paradigma dei "due popoli, due stati", avevano aperto una nuova strada avevano costretto alcuni Paesi arabi, soprattutto le monarchie del Golfo, a misurarsi con il riconoscimento di Israele e a parlare con gli israeliani. A questo punto, però, va chiesto di essere conseguente, perché l'apertura di credito che è stata data ha bisogno di essere sostenuta. E chi, se non gli Stati Uniti, possono aprire questa nuova fase?

Non a caso, l'ala sinistra del suo partito, con in testa giovani donne progressiste e democratiche come Ocasio-Cortez, lo richiama a essere coerente, perché

Lei ha misurato con mano la difficoltà di costruire anche una sola posizione comune: il difficile compito di Borrell, nel momento in cui si confronta con il blocco orientale di Paesi come l'Ungheria e la Polonia, che non si

forte ha bisogno di più coraggio: non basta il coordinamento della politica estera e della difesa, ma abbiamo bisogno di investire di più sull'Europa. Per affrontare le grandi sfide internazionali serve un'Europa politica unita, con un'unica politica estera e un'unica politica di difesa. Dobbiamo avere più coraggio.

ringraziamo per la sua informativa, che abbiamo apprezzato, e per aver accolto la sollecitazione, portata avanti dal nostro Gruppo, per discutere di ciò che sta avvenendo in queste settimane in Palestina. Lo abbiamo fatto, in primo luogo, per sollecitare e sostenere un'iniziativa internazionale per l'immediato cessate il fuoco. Il prezzo che stanno pagando i civili e i bambini è troppo alto e non può essere che inaccettabile per tutta la comunità internazionale. Il poco tempo a disposizione impone di partire da elementi di verità, di verità, che nella narrazione generale - bisogna riconoscerlo - è sostanzialmente oscurata. Troppe parole di circostanza si sono sentite in questi giorni. Occorre capire il contesto, che ci spieghi cosa sta effettivamente succedendo. Non basta condannare le azioni criminali e violente di Hamas, né affermare che la difesa di Israele, senza mai dimenticare la disparità delle sue forze rispetto ai palestinesi, non può arrivare a colpire i civili, i bambini, gli ospedali e l'informazione internazionale. C'è bisogno, oltre all'immediato cessate il fuoco, di una nuova iniziativa internazionale, che superi l'inerzia colpevole di questi anni e, con coraggio e determinazione, faccia un'operazione di verità, non rimuovendo la questione palestinese, come purtroppo si è fatto in questi anni. Diversamente - lo voglio dire con chiarezza, come hanno fatto già altri colleghi, che ho apprezzato - l'affermazione "due popoli, due Stati" suona come un'inutile e vuota retorica. Sottolineo

per la capacità di stimolare il dialogo di pace e il confronto tra palestinesi e israeliani. un valore che non dobbiamo disperdere e ho apprezzato per questo la sua comunicazione, signor si è via via lasciato che prendessero piede gli estremismi, sia nel popolo palestinese, sia nel popolo israeliano, israeliano, che si sono alimentati nella ricerca, di fatto, non di una soluzione pacifica, bensì di un'assurda soluzione finale. Così si è alimentato, negli anni, un drammatico circuito vizioso. Israele si sente sempre più insicuro, il popolo palestinese vive, di fatto, da decenni, una situazione di occupazione militare, mentre l'altra parte, quella degli arabi israeliani, vive una situazione di cittadinanza subordinata nello Stato di Israele, che li tratta come ospiti, con diritti differenti. In questi anni, si è lasciata mano libera alla politica di occupazione dei territori palestinesi, senza che nessuno intervenisse. Nessuno può accettare che sia messa in discussione la sicurezza di Israele, ma dobbiamo chiederci se sia stato giusto lasciare che le risoluzioni dell'ONU venissero così platealmente ignorate. Tutto ciò a cosa ha portato? Come si è arrivati al punto che l'islamismo di Hamas e il ruolo di Erdogan abbiano assunto un ampio consenso nel mondo arabo? Un punto di rottura drammatico è stato sicuramente il riconoscimento da parte di Trump di Gerusalemme come capitale dello Stato israeliano. Forse non capiamo bene la portata di questa scelta, sciagurata e simbolica, con un peso enorme in quel territorio, che ha messo ulteriormente e pesantemente in crisi la situazione in Medio Oriente, stracciando ancora una volta le specifiche risoluzioni dell'ONU. Gli scontri dei giorni passati sulla spianata delle moschee ad opera degli arabi israeliani - arabi israeliani, cittadini israeliani - sono il frutto - perché nasconderlo? - di scelte unilaterali del Governo Netanyahu, come la minaccia di sfratto di una ventina famiglie nel quartiere di Gerusalemme Est, basato su una causa legale vecchia di cento anni. Il problema però, evidentemente, non era la causa legale. Si parla dello Stato palestinese, ma procede la colonizzazione dei territori che sostanzialmente non hanno più un'unità amministrativa. Tutto ciò

che, con la sua follia e violenza, è paradossalmente il migliore amico dell'estrema destra israeliana. Del resto, è evidente che Hamas e l'estrema destra israeliana si tengono e che drammaticamente il loro ruolo è tutto a discapito sia della sicurezza del Popolo israeliano sia della causa del popolo palestinese e del processo di pace. Lo dimostra il fatto che questi avvenimenti hanno già prodotto due effetti molto negativi: il 22 maggio dovevano tenersi, dopo quindici anni, come giustamente ha ricordato lei, le elezioni in Palestina, nelle quali si stava profilando la sconfitta di Hamas e la nascita di una nuova dirigenza palestinese, capace forse di portare avanti il dialogo in Israele. Dall'altra parte, in Israele, dopo quattro elezioni politiche in due anni, si stava formando una coalizione che avrebbe potuto raggiungere la maggioranza parlamentare grazie anche ai quattro voti parlamentari del Partito arabo israeliano. Non sarà un caso che è successo tutto questo, un evento che avrebbe aperto una fase nuova nel rapporto con gli arabi israeliani e nella politica di Israele. Dopo la crisi, queste possibilità sono svanite. Questa spirale di violenza va interrotta ora attraverso l'iniziativa internazionale, un nuovo ruolo degli Stati Uniti e dell'Europa, un ruolo meno timido rispetto a quello di questi anni, particolarmente negli Stati Uniti. Ciò che è avvenuto sui pescherecci italiani è inconcepibile. Non è la prima volta. Condividiamo le cose che ha detto sulla Libia e sulla e sulla questione della pesca; occorre però, signor Ministro, come da tempo chiediamo, una scelta. Il rapporto con la guardia costiera Libica va risolto va ridiscusso il rapporto col Governo libico, perché siamo di fronte, come i tanti rapporti internazionali ci dicono, a una serie di comportamenti di costante e inaccettabile violazione dei diritti umani. Infine, signor Ministro, una il Senato ha chiesto con una mozione di dare la cittadinanza italiana a Zaky. Quali iniziative prendiamo?

per le sue parole nette ed inequivocabili di condanna rispetto ad Hamas come organizzazione terroristica. Se la comunità internazionale non ha il coraggio di mettere al bando questa organizzazione, purtroppo la pace in quella terra sarà molto difficile raggiungerla. un certo tipo di intervento, ma ascoltandone alcuni recenti interventi vorrei suggerire una lettura un po' meno pregiudizievole, meno ricca di luoghi comuni. Israele nasce, come lei ben sa, nel 1948 da da una determinazione delle Nazioni Unite. Quella terra era divisa in due Stati, lo Stato di Palestina e lo Stato di Israele. I palestinesi non hanno accettato quella risoluzione, soprattutto i Paesi del Golfo Persico. Israele l'ha accettata ed è diventato uno Stato, ha coltivato e cresciuto tutti i fondamentali di una democrazia. Come lei ben sa, chi governa un territorio deve garantire due principi fondamentali: la pace per il suo popolo e la prosperità. In tutti questi anni Israele non ha mai posto in essere alcun atto di aggressione nei Paesi confinanti. Tutta la storia recente di questo Stato ci racconta che ha sempre subito aggressioni militari da parte dei Paesi confinanti. Vorrei ricordarne alcune. La più importante fu la guerra dei sei giorni. In quel caso non è Israele che ha attaccato, ma ha subito un attacco;

come ho sentito dire da qualche collega che mi ha preceduto, che Israele non ama la pace: Israele è cultrice della pace, perché senza la pace non può garantire la prosperità al suo popolo. Così è andata avanti con i trattati di Oslo e quindi con i trattati bilaterali con la Giordania e con altri Paesi. Non vorrei ricordare tutti i trattati. Mi dispiace che su Trump qualcuno abbia glissato, perché Trump ha avuto un merito: dopo trent'anni di totale accantonamento, con ha detto il presidente Casini, della politica sul Medio Oriente, qualcuno ci ha messo le mani ed ha raggiunto un altro accordo di normalizzazione con Paesi arabi, penso al Bahrein e penso agli Emirati arabi. Attenzione, quindi, perché è vero che molte dinamiche sono frutto di politiche domestiche, ricordo semplicemente che il Medio Oriente è un palcoscenico internazionale, molti sfruttano la Palestina come palcoscenico internazionale ed è uno scontro tutto interno all'Islam, che da anni si perpetra in diversi luoghi tra sunniti (che si conformano alla Sunna) e sciiti e questo rischia di diventare, purtroppo, un elemento disgregante. Difficilmente si può aggiungere la pace se non comprendiamo questi elementi. Ricordo ai colleghi che Israele popolata da 8,3 milioni di persone, forse pochi lo sanno. Io sono cristiano, sono nato in quella terra e non credo di avere meno diritti rispetto agli ebrei di quella terra, nella maniera più assoluta, ricordo a tutti quanti noi che 1,3 milioni di israeliani sono arabi di fede musulmana islamica e non credo che abbiano diritti inferiori.

e la stragrande maggioranza rispetta le regole democratiche, rispetta lo Stato di Israele. Il suggerimento, quindi, è di non cadere nei luoghi comuni. Quella è una democrazia, al netto delle politiche domestiche che posso anche condividere, ma non possiamo mettere sullo stesso piano le varie dinamiche di quel territorio. Vorrei inoltre soffermarmi su

reagire in modo proporzionato? E chi determina qual è la proporzione? Questo è un tema su cui auspico che ci sia un dibattito più scevro da polemiche e da pregiudizi. Tutti noi speriamo che lì nasca la pace, ma attraverso il riconoscimento dello Stato d'Israele, perché ho difficoltà a immaginare che uno Stato possa tollerare di sedersi a un tavolo con un altro che sostiene che non dovrebbe esistere. Israele, nella sua storia

Un ultimo suggerimento, signor Ministro: sulla Libia, io la ringrazio per la sua capacità di moderazione e di prudenza, tipica della diplomazia italiana. Va bene essere equi e vicini, come diceva un dotto democratico cristiano, ma talvolta bisogna anche scegliere, perché, se non scegliamo, rischiamo che nasca la palude. E nella palude succede quello che sta accadendo in questo momento in Israele.

del signor Ministro un altrettanto importante problema che affligge l'Italia da molto tempo. Nonostante il nostro puntuale conformarci alle molteplici leggi europee ed internazionali, non sempre vi è stata reciprocità con le altre Nazioni. Riprendo i fatti che lei ha citato poc'anzi, avvenuti tutti in acque internazionali e che hanno visto protagoniste la Libia, la Tunisia, la Turchia la guardia costiera libica, che ha sequestrato un peschereccio italiano col suo equipaggio. In altra occasione, il comandante di una motonave italiana è stato ferito da colpi di arma da fuoco da un'imbarcazione libica: quasi una beffa, se si pensa che era una di quelle donate dall'Italia alla Libia. Se non fosse prontamente intervenuta la nostra Marina militare, questo episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In Italia non si sono mai fermati i flussi migratori dalla rotta balcanica, come pure le migliaia di immigrati che salpano dalle coste turche, in arrivo anche in questi giorni su barchini, barche a vela e imbarcazioni di fortuna. È importante, però, chiarire una contraddizione in atto. Se il nostro Ministro dell'interno, per difendere i nostri confini europei e la redistribuzione delle persone che giungono nel nostro Paese, chiede la concreta ed efficace solidarietà dell'Europa, come può, poi, una nave tedesca raccogliere 400 persone in acque libiche e maltesi e dirottarle unicamente in Italia, perché lo Stato maltese si rifiuta di accoglierli? *(Applausi)*. Le norme che regolamentano le acque internazionali indicano che queste persone possano chiedere asilo alla Nazione di bandiera della nave che le ha tratte in salvo. Invece, la domanda d'asilo viene da loro chiesta solo dopo lo sbarco sul suolo italiano. L'imminente arrivo della bella stagione comporterà un incremento di questo fenomeno. Se da gennaio ad oggi contiamo più di 13.000 immigrati, il livello di preoccupazione si farà ancora più alto. Sembrano pronti a partire già in 65.000. Inoltre, l'esito di recenti indagini della magistratura ha riscontrato comportamenti illeciti fra organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani, ben lungi dal potersi considerare aiuti. Lo strumento del soccorso così impostato, senza nessuna regola anche di identificazione, ha comportato lo sbarco di soggetti dediti alla delinquenza. Penso di non dovermi soffermare su particolari episodi: basta guardare i quotidiani che riportano costanti atti di violenze ai danni di donne, bambini e uomini italiani, del tutto inconsapevoli di diventare oggetto di barbarie. Spostandoci, poi, sotto il profilo economico, è bene ricordare il sostenuto indebitamento di bilancio (200 miliardi di scostamento) il ricorso ad altrettanto indebitamento europeo, oltre 200 miliardi sul PNRR che abbiamo in quest'Aula approvato. Le nostre famiglie non sono in grado di garantirsi un lavoro, di pagarsi il mutuo, di pensare al futuro dei propri figli. Questa è forse la risposta alla grave crisi demografica italiana e agli infruttuosi incentivi sulla natalità? I cittadini sono allarmati, non comprendono perché lo Stato non riesca a dare risposte più incisive, sentono la mancanza di una giusta tutela sia giuridica che economica, pur comprendendo la necessità di non essere indifferenti nei confronti di chi è realmente bisognoso. Mi si permetta una citazione importante, forte ed antica, ma quanto mai attuale: Cristo, Platone ammoniva gli ateniesi dicendo loro: «quando il cittadino accetta che chiunque gli capiti in casa possa acquistarvi gli stessi diritti di chi l'ha costruita e ci è nato, quando i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi in nome di una libertà che divora e corrompe ogni regola, così muore la democrazia: per abuso di sé stessa. E, prima che nel sangue, nel ridicolo.

stasera ho messo i bambini a dormire nella nostra camera da letto, in modo che quando moriremo, moriremo insieme e nessuno vivrà per piangere la perdita l'uno dell'altro. Queste sono le parole di una mamma di Gaza, una mamma rassegnata alla morte, una madre che vede limpidamente il destino della sua famiglia segnato dall'orrore della guerra. Moriremo tutti insieme, così nessuno dovrà piangere l'altro. Un pensiero colmo d'amore nel mezzo di una guerra. Odio e violenza dove porteranno? Servono dialogo e perdono. Queste sono le parole di Papa Francesco. Questa guerra ha prodotto l'ennesima strage degli innocenti: i morti sono più di 250, di cui 12 dal lato israeliano e 240 dal lato palestinese, ma si può mai fare la contabilità dei morti?

per essere nati in un fazzoletto di terra conteso da uomini potenti che dicono di volere la pace, ma continuano a fare la guerra. I morti sono morti. Mi hanno insegnato che le vittime non hanno colore e che la violenza va condannata sempre, a prescindere da chi vi ricorre. Amnesty international parla di crimini di guerra, non solo per l'indiscriminato lancio di razzi da Gaza, ma anche per i bombardamenti israeliani sulla striscia che hanno colpito senza preavviso molti edifici civili, compresi due che non sembrano essere obiettivi militari, ovvero la torre che ospitava la sede di Al Jazeera e l'agenzia di stampa Associated Press, e l'unico laboratorio di analisi di tamponi Covid presente nella striscia di Gaza. striscia di Gaza la situazione legata alla pandemia è già drammatica. Ad aprile 2021 il 60 per cento degli israeliani risultano vaccinati, contro solo l'1 per cento dei palestinesi.

Medici senza frontiere parla di una goccia in mezzo al mare; Save the children ha dichiarato che nell'ultima settimana a Gaza sono state distrutte o fortemente danneggiate 50 scuole. Che futuro si garantisce ai bambini se le scuole vengono distrutte? Nonostante l'evidente sproporzione di forze, le vittime di questa situazione sono entrambi i popoli che subiscono le conseguenze delle azioni di chi vuole la guerra. Chi la vuole non è mai il popolo, che la guerra la subisce, ma chi usa la guerra per mostrare i muscoli e conservare o prendere il potere. Da entrambi i lati la guerra è usata per biechi giochi di potere. Quattro elezioni parlamentari in due anni, da un lato, e nessuna elezione dal 2006, dall'altro, testimoniano, infatti, una situazione di stallo impressionante, che ha portato all'inasprimento delle posizioni e alla strumentale riesplosione delle tensioni. La guerra fa schifo! La guerra dovrebbe diventare un tabù, come dice un sacerdote che conosco. La comunità internazionale ha il dovere di agire, di sedare le lotte e far cessare il fuoco, questa volta in maniera definitiva e per sempre. Razzi, mortai, missili e tutti gli strumenti di guerra devono essere dismessi, a partire da quell'area. La pace non si fa con la guerra. Deve essere ripristinato il rispetto del diritto internazionale e di tutte le risoluzioni dell'ONU. I diritti umani non sono negoziabili; non lo è il diritto a vivere serenamente nelle proprie case e neanche il diritto a esistere, sia quello dei palestinesi che quello di Israele. In una tragedia, come quella che vive il Medio Oriente, bisogna essere uniti nel gridare «cessate il fuoco». Dopo bisognerà agire per riannodare il dialogo tra le parti e arrivare all'unica soluzione logica: quella di due Stati secondo i confini indicati nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in particolare la n. 2334 del 2016, che sancisce l'illegalità di tutti gli insediamenti israeliani stabiliti nei territori occupati in Cisgiordania e in Gerusalemme Est. Annessioni, demolizioni e sfratti generano frustrazione e contribuiscono alla violenza e per questo vanno condannati, senza alcun timore. Nel 2017 l'allora presidente Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale indivisa dello Stato di Israele. Papa Francesco ha subito detto che Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani e ha una vocazione speciale alla pace, di cui bisogna rispettare lo *status quo*. Il piano Trump del 2020 ha poi legittimato tutte le annessioni territoriali israeliane, in aperto contrasto con le risoluzioni dell'ONU. Il cambio radicale della politica americana dell'era Trump non ha prodotto gli effetti di pacificare l'area, anzi, ne ha esaltato le contrapposizioni, destabilizzando equilibri già precari, non solo nei territori palestinesi, ma anche in Israele, dove il 21 per cento della popolazione è di origine araba. È ora che gli Stati Uniti, per il bene del loro storico alleato, tornino a svolgere un ruolo di mediazione per fermare il conflitto e riavviare il processo di pace. Per questo è fondamentale anche il contributo dell'Italia e dell'Europa. Crediamo fortemente che la Presidenza italiana del G20 sia l'occasione per il nostro Paese per promuovere un approccio laico alla questione israelo-palestinese. Proprio in quest'ottica, una volta che le bombe, i missili e i razzi avranno smesso di cadere, penso sia doveroso che il Parlamento italiano si esprima a favore del riconoscimento dello Stato palestinese *(Applausi)*, nei confini precedenti l'occupazione del 1967, con Gerusalemme capitale condivisa, così come previsto dalle risoluzioni ONU e come hanno già fatto 139 Stati, compreso il Vaticano. Già nella scorsa legislatura il MoVimento 5 Stelle si è espresso sul tema e nel 2019, con la mozione a prima firma del collega Gianluca Ferrara, abbiamo chiesto al Governo di riconoscere lo Stato di Palestina e di proporre che facciano altrettanto tutti i Paesi dell'Unione europea. Sarebbe un importantissimo contributo a una pace giusta e duratura, basata sul rispetto del diritto internazionale e delle legittime aspirazioni di entrambi i popoli a vivere in pace e in sicurezza. In conclusione, un accenno sulla Libia; la sua stabilizzazione e normalizzazione sono una priorità assoluta per il nostro Paese, per il ruolo che ha avuto l'Italia in quell'area e, in particolare, per il settore della pesca e per quello energetico. Un pensiero va ai nostri pescatori di Mazara del Vallo, che spesso si sono trovati a lavorare in acque pericolose. Il nostro Paese deve continuare a lavorare, anche se il percorso è ancora lungo ed è reso difficile dall'influenza e dagli interessi di altri Paesi. Anche per questo ritengo che tutti abbiamo il dovere di tornare a impegnarci per chiudere definitivamente il vaso di Pandora scoperchiato con il folle intervento armato del 2011. Concludendo e tornando al Medio Oriente, voglio chiudere con le parole di Franco Battiato, grande poeta italiano scomparso ieri. In un passaggio di una sua canzone diceva: «Com'è misera la vita negli abusi di potere». È bene che ce lo ricordiamo tutti. *(Applausi)*.

Signor Presidente, oggi abbiamo esaminato diverse relazioni sulla base dell'articolo 68 della Costituzione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni, tra cui anche la mia. Anzi, colgo l'occasione per ribadire che non ho votato a favore *(Applausi)*, come ha affermato un collega. L'Assemblea ha votato prendendosi la responsabilità politica verso i cittadini e verso i propri elettori mettendoci, come si suol dire, la faccia. Durante la discussione, però, mi sono venuti in mente anche gli articoli 54 e 64 della che i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, mentre l'articolo 64 enuncia l'autonomia delle due Camere. Allora, dov'è finito l'articolo 54 se è normale annullare una delibera del Consiglio di Presidenza che sospendeva i vitalizi agli ex senatori E dov'è finito l'articolo 64 se un organo giurisdizionale interno, formato da politici non interamente espressione del popolo può annullare, come è successo ieri sera, una delibera del Consiglio di Presidenza in cui sono rappresentate tutte le forze politiche? Vorrei andare oltre le frasi "vitalizi sì" o "vitalizi no", perché mi rendo conto che se non si sciolgono alcuni nodi sulla disciplina e l'onore dei rappresentanti del popolo, il Senato rischia di dare uno schiaffo ai cittadini che in piena pandemia non riescono ad arrivare a fine mese. Invito quindi tutti i colleghi a una discussione in Aula, perché solo così i cittadini potranno capire da che parte sta la politica.

è il nono anniversario del terremoto dell'Emilia. Alle ore 4,03 del 20 maggio 2012, un severo scuotimento del suolo colse di sorpresa l'Emilia; in realtà, nulla di sorprendente, se non l'ignoranza e la negligenza, ancora oggi imperanti in tema di rischio sismico. Lì il terremoto aveva già duramente colpito in passato, ma si dimentica; ricordare serve al futuro. La ben nota compressione della placca adriatica verso l'Europa ha riattivato due ben note faglie inverse che hanno originato i terremoti del 20 e 29 maggio 2012, di magnitudo 5.9 e 5.8, e di intensità fino all'ottavo grado della Questi terremoti hanno duramente colpito la bassa modenese: 1.000 chilometri quadrati, 230.000 persone coinvolte. Carpi, Cavezzo, Finale, Medolla, Mirandola, Novi e molti altri Comuni hanno subito ingentissimi danni: colpiti centri storici, edifici rurali e capannoni; ventisette vittime, per lo più dipendenti di aziende distrutte; colpiti scuole, ospedali e chiese; danni per oltre 13 miliardi di euro. Buona è stata invece la risposta degli edifici costruiti recentemente in calcestruzzo. è l'ennesima conferma che, riducendo la vulnerabilità, si minimizza il rischio sismico. La normativa vigente per quest'area contempla che le nuove costruzioni non debbano collassare se sollecitate da una accelerazione orizzontale di picco al suolo (PGA) fino al 15 per cento dell'accelerazione di gravità, qui statisticamente prevista con tempi di ritorno di 475 anni, al netto dei fenomeni locali di amplificazione del moto. In realtà, a Mirandola si registrò una PGA del 30 per cento, ossia il doppio, prevista con un tempo di ritorno di 2.475 anni. Costruire e adeguare con questo limite più cautelativo che sto proponendo in decreti e disegni di legge avrebbe impedito crolli e morti. Nel terremoto in oggetto molti danni sono poi stati provocati da effetti geologici secondari, quali la liquefazione dei suoli. Tali effetti possono essere prevenuti con studi di microzonazione sismica, che consente un'adeguata pianificazione. Occorre Occorre ad ogni costo investire in conoscenza e prevenzione. Prevenire il rischio sismico costa dieci volte di meno che ricostruire ed evita tragedie.

il 28 aprile di quest'anno la gioielleria del signor Roggero è stata oggetto di una tentata rapina finita nel sangue. Il signor Roggero ha reagito, ha ferito mortalmente due rapinatori e in maniera meno grave un terzo ed è oggi accusato di eccesso di legittima difesa. Ma cosa vuol dire eccesso di legittima difesa? I tre sono entrati in negozio armati di coltello e rivoltella, risultata poi un giocattolo a cui avevano tolto il tappino rosso che la identificava come finta; hanno tirato un pugno alla moglie e immobilizzato la figlia con fascette da elettricista, si sono fatti consegnare dei gioielli e quando ha potuto il signor Mario ha reagito. Ma cosa può spingere un onesto uomo di sessantasei anni, che non ha mai avuto problemi con la legge, a sparare? Ve lo dico io: la paura. Paura per sé e soprattutto per la propria famiglia. Sì, perché il signor Roggero è un esperto in gioielli e non un perito balistico, perché nel 2011 era già stato rapinato e brutalmente malmenato da malviventi e solo dopo questo fatto aveva acquistato una pistola. E poi, coltello e pugno erano veri, tremendamente veri. Se dobbiamo identificare delle vittime, queste non sono sicuramente i rapinatori: due delinquenti con precedenti penali che volevano fare il salto di qualità, muniti di pistola giocattolo perché consapevoli del fatto che, in caso di arresto, non avrebbero avuto aggravanti. Persone che chissà quante altre volte avevano terrorizzato per rapina brava gente, con armi vere o finte che fossero, e che ora volevano fare, appunto, il salto di qualità. Sono vittime il signor Mario e la sua famiglia. Credo sinceramente che attualmente abbia dei seri problemi la sera ad addormentarsi, perché uccidere qualcuno sconvolge le persone per bene. La fortuna ha voluto che i due fossero colpiti al torace e non alle spalle, altrimenti per lui sarebbe iniziato un interminabile calvario giudiziario e mediatico. Conosco bene le emozioni che la famiglia Roggero può aver provato in quanto sono una loro collega; so bene l'agitazione e l'attenzione che ognuno di noi prova quotidianamente nei due momenti critici dell'apertura e della chiusura del negozio, oppure quando entra un cliente e capisci che è molto più interessato al tipo di impianto d'allarme che alla merce che ti ha chiesto di vedere. E soprattutto, so bene cosa si prova quando puntano la pistola alla testa di qualcuno a cui vuoi bene. Nel mio caso le hanno puntate, in due diverse tentate rapine, a mio nonno e mia nonna. Non oso pensare come avrei reagito se a loro posto ci fosse stata mia figlia. Per concludere, dal mio punto di vista il signor Roggero è un eroe. *(Applausi)*. Ha semplicemente difeso famiglia e proprietà dall'intrusione di qualcuno che scientemente era entrato con intenti ostili e violenti. Altro che processo, meriterebbe un plauso. Chi decide di violare la proprietà altrui con intenti malvagi deve mettere in conto di poterne uscire male o, a volte, di non poterne uscire. Siamo dalla parte del signor Mario e di tutti coloro che si sono trovati o si troveranno nella sua situazione, perché la difesa deve essere sempre legittima.

sono cinque anni che Pannella ha trovato un modo diverso per essere presente nella politica italiana e certo ci manca in questi cinque anni la sua presenza fisica, che era irruente, metteva il corpo nelle sue azioni e metteva la vita per dare la forza agli altri di fare ciò di cui avevano bisogno. bisogno. Però, in questi cinque anni, sono tanti i temi che Marco Pannella ha provato a sottolineare nel dibattito politico e su cui ci sarebbe stato prezioso il tuo punto di vista. Proviamo, a fare di questa sua mancanza una presenza. Penso allo sterminio per fame, a quanto è importante oggi nella dinamica delle migrazioni, invece che raccontarla in maniera semplicistica in altro modo. Penso al dibattito che abbiamo appena avuto su Israele e Palestina, a quella proposta lungimirante di uno Stato bi-nazionale che garantisca i diritti di cittadinanza di tutti e che sia garantito a sua volta dall'Unione europea. Proprio sull'Europa, in questo momento che è in corso la conferenza sull'Unione europea, pensare a un'Europa che sia più larga, più grande, più federale, che superi la forma degli Stati nazionali. E ancora, la giustizia con la riforma che questo Governo vuole portare avanti, le carceri: sono tanti i temi, e su tutti il rapporto con l'altro, il metodo non violento, l'idea del dialogo, la funzione del Parlamento, la centralità della politica. Ecco, di tutti questi ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore. L'ultima battaglia di Marco Pannella fu quella per il diritto alla conoscenza, che è alla base della democrazia. Proprio tra pochi giorni, il prossimo venerdì, nella Commissione cultura dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa approveremo il mio rapporto sul diritto alla conoscenza, che inizierà il percorso - che si concluderà nel mese di giugno, dopo due anni - per far diventare questo un nuovo diritto umano. Credo che, a cinque anni da questo cambiamento del modo di essere presente di Marco Pannella nella politica italiana, questo sia un piccolo traguardo che consegniamo per

Grazie